in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, è convertito in legge con le modificazioni

Signor Presidente, onorevoli colleghi. come già avevo espresso nel mio intervento alla Camera dei deputati, questo testo normativo si inserisce in un disegno ampio e complessivo del Governo Meloni, nella convinzione che il fenomeno epocale dei flussi migratori vada governato dallo Stato e non subìto, perché questo è l'unico modo di poter coniugare i diritti di chi cerca un futuro migliore nel nostro Paese con il contrasto agli interessi di organizzazioni criminali transnazionali che lucrano guadagni enormi in assoluto spregio alla vita di queste persone. Questo è il fine principale. Trovo irricevibili e anche offensive le parole di chi ci ha mosso accuse di razzismo e crudeltà: i buoni, sempre pronti a dare lezioni di umanità, coloro che in questi anni hanno sostenuto l'immigrazione indiscriminata e senza regole, senza proporre alcuna soluzione alternativa a quella della redistribuzione, di cui conosciamo bene i risultati. È proprio la politica dei porti aperti quella che porta migliaia di persone ad affrontare i rischi delle traversate nel Mediterraneo su carrette sgangherate, affidandosi a trafficanti senza scrupoli.

Sono costretti a sopravvivere come fantasmi ai margini delle nostre città, a commettere reati per procurarsi da vivere, a diventare manovalanza per le organizzazioni criminali o schiavi per i caporali, che li sfruttano come forza lavoro a basso costo e senza diritti, a beneficio di imprenditori senza scrupoli. quante inchieste ci hanno svelato qual è il grande *business* che ruota attorno all'accoglienza, quante cooperative trattano questi uomini e queste donne come merce da rimborso, senza garantire i diritti - se non per qualcuno il diritto all'eleganza - senza garantire salute, senza garantire dignità. Più migranti arrivano, più si gonfiano le tasche di sfruttatori ad ogni livello, dalla partenza all'accoglienza, allo sfruttamento lavorativo. È allora forse il momento di uscire dall'ipocrisia. Chi è il razzista, mi chiedo? Chi per anni ha creato questa realtà di emarginazione, che crea condizioni di insicurezza nelle nostre comunità e quindi alimenta la paura e il fenomeno del razzismo. Certo non chi, come noi, vuole stabilire regole che diano risposte a queste persone, che che noi vogliamo arrivino in Italia, perché ne abbiamo bisogno certamente, perché rispondono alle richieste di forza lavoro del nostro sistema economico e produttivo e spesso alle necessità delle nostre famiglie, che hanno bisogno di aiuto per assistere i più fragili, ma questo deve avvenire in un contesto di legalità, dignità, diritti e integrazione sociale. Questo Governo sta lavorando per garantire una migrazione legale con regole certe, semplici e chiare, con l'obiettivo di consentire un numero ampio di ingressi regolari sostenibili, in modo da assicurare l'inserimento lavorativo degli stranieri che che possono dare il loro contributo alla nostra comunità solo se possono avere un lavoro sicuro, tutelato e ben pagato e non se utilizzati per creare una competizione al ribasso sul valore del lavoro e sui diritti. Le politiche messe in campo dal Governo, incentrate sulla lotta all'immigrazione irregolare e sulla promozione di canali di immigrazione legale stanno dando i propri frutti. Dall'inizio dell'anno al 3 dicembre sono giunti sulle nostre coste 63.537 migranti,

ma nessuno prima d'ora ha mai fatto qualcosa per cambiarla, se non sostituire, di fatto, le quote d'ingresso legali con quelle provenienti dall'immigrazione irregolare e incontrollata. Questo Governo è convinto che le migrazioni debbano essere gestite nella direzione di una reale integrazione, che significa dare a questi migranti l'opportunità di essere membri attivi della nostra società, innanzitutto attraverso l'inserimento lavorativo, che, come dicevo, rappresenta anche un'opportunità di crescita economica per le nostre aziende che in tanti settori che soffrono la carenza di manodopera. È attraverso il lavoro che il migrante può sentirsi davvero parte integrante e dare il contributo attivo alla comunità, stabilendo relazioni, apprendendo la lingua, comprendendo meglio la cultura. Questo processo di integrazione è fondamentale per prevenire fenomeni di isolamento sociale e discriminazione, ma anche situazioni di grande insicurezza in tanti territori. Noi vogliamo fare in modo che chi è costretto a lasciare il proprio Paese d'origine per lasciarsi alle spalle persecuzioni, violazioni di diritti, ma anche chi vuole migliorare la propria condizione - e noi continuiamo e continueremo a lavorare perché perché emigrare sia una scelta e non una disperata costrizione - comprenda la necessità di farlo accedendo ai canali legali e sicuri, anziché affidando la propria vita ai trafficanti. È questo l'obiettivo del lavoro che il Governo sta portando avanti di cui questo provvedimento è parte integrante. Esso si muove su tre direttrici. La prima è la lotta all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, anche attraverso una più stretta cooperazione internazionale. Ricordo ancora una volta i numeri del traffico di migranti, che genera un giro d'affari annuo che oscilla tra i 4,7 e i 6 miliardi di euro all'anno; un *business* criminale che ha raggiunto, per volumi di denaro, volumi di denaro, il traffico di droga o quello di armi. Negli ultimi due anni le nostre Forze di polizia hanno arrestato 470 scafisti. Grazie alla cooperazione con le autorità libiche e tunisine, abbiamo bloccato quest'anno 96.736 partenze di migranti irregolari, che si aggiungono alle 93.511 partenze bloccate nel 2023. La seconda direttrice è la promozione di canali di immigrazione legali e sicuri, ragione per cui abbiamo favorito una migliore programmazione di ingressi regolari, stabilendo nel prossimo triennio un flusso regolare di 450.000 migranti. numeri di gran lunga superiori a quelli del passato, quando le quote erano sempre assorbite dall'immigrazione clandestina. La terza direttrice, più a lungo termine, è la volontà di incidere, attraverso il famoso Piano Mattei, sulle cause di fondo dei flussi migratori, promuovendo a livello internazionale il sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi di partenza e progettando investimenti a medio e lungo termine per garantire il diritto a non emigrare, a non costringere migliaia di giovani a recidere le proprie radici per costruirsi un futuro lontano dalla propria terra; un diritto al quale pochi sembrano dimostrarsi attenti e sensibili, perché non risponde a quella visione ideologica mondialista tanto cara alla grande finanza speculativa che nega le identità nazionali e il valore dei legami dei legami comunitari. La linea del Governo prosegue dunque nell'ottica di concorrere al consolidamento della stabilità politica, economica e sociale dei Paesi di partenza. Evidenzio, al riguardo, che proprio in questi giorni il Ministro dell'istruzione e del merito ha effettuato una missione in Algeria, durante la quale sono stati firmati due *memorandum* d'intesa destinati a rafforzare la collaborazione italo-algerina nei campi dell'educazione e della formazione tecnico-professionale e tecnologica. Ci avete accusato di tante cose, tra cui di confusione e di avere emanato 8 provvedimenti in materia di immigrazione in due anni, ma ritengo che questo esprima la nostra grande determinazione a dare risposte efficaci ad una materia complessa e in continua evoluzione. Ricordo che questo provvedimento nasce proprio dalla necessità di prevedere dei correttivi a seguito del monitoraggio degli effetti dei decreti flussi per il triennio 2023-2025 effettuato da questo Governo, che ha portato all'individuazione di gravi anomalie, che hanno fatto emergere l'utilizzo illecito l'utilizzo illecito dei flussi lavorativi da parte dei gruppi criminali, e sul quale si stanno sovrapponendo anche decisioni giurisdizionali che hanno fatto emergere criticità, a nostro avviso, di carattere interpretativo, alle quali abbiamo ritenuto di dover dare una risposta. Abbiamo parlato dei Paesi sicuri. Questo aspetto nel dibattito di ieri, è stato fatto emergere da molti Gruppi. Il provvedimento include l'aggiornamento della lista dei Paesi sicuri per il rimpatrio degli immigrati irregolari, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, rendendo

frutto di un complesso lavoro e procedimento di carattere politico-amministrativo, è di competenza degli Stati membri, come riaffermato anche dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. È una direttiva europea (la n. 32 del 26 giugno 2013), infatti, a introdurre le procedure accelerate di frontiera, con la previsione che uno dei requisiti per l'applicazione sia che il migrante irregolare provenga da un Paese sicuro, senza tuttavia definire alcuna lista di Paesi sicuri e demandando dunque questa competenza agli Stati membri. Nello specifico, è stato richiamato l'articolo 36, che esplicita il concetto di Paese di origine sicuro e precisa che un Paese terzo può essere considerato Paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se questi ha cittadinanza di quel Paese ovvero è un apolide che in precedenza vi soggiornava abitualmente e non ha invocato gravi motivi per ritenere quello non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95 prevede inoltre - questo lo voglio sottolineare - che siano gli Stati membri a stabilire nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di Paese sicuro. L'articolo 37 della direttiva dispone, a sua volta, che gli Stati membri abbiano la possibilità di mantenere in vigore e introdurre una normativa che consenta di designare a livello

detta un elenco puntuale dei Paesi di origine sicuri, tali nell'interezza del loro territorio, da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge. Esso inoltre prevede, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, un'informativa annuale del Governo mediante una relazione che viene trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. La nuova disposizione enumera essa stessa il novero dei Paesi di origine da ritenersi sicuri. L'individuazione dei Paesi sicuri avviene quindi… *(Brusìo)*. Presidente, è veramente complicato

L'individuazione dei Paesi sicuri avviene quindi in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea ed è frutto di un procedimento complesso di carattere politico e amministrativo, che tiene conto di informazioni, in alcuni casi anche abbastanza riservate provenienti proprio dall'*intelligence*, e di valutazioni politiche, legali e sociali, che richiedono competenze specialistiche che il singolo magistrato non può avere. Non voglio fare in questa sede considerazioni sulle prese di posizione di alcuni tra i magistrati che non hanno convalidato i trattenimenti dei migranti. ho sempre avuto grande rispetto della magistratura; non cadrò mai nella trappola di chi fa una narrazione e un racconto della politica contro la magistratura. Penso solo che l'interpretazione della sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia dell'Unione europea fatta dai giudici italiani nei provvedimenti di mancata convalida dei trattenimenti dei migranti nei centri in Albania, che non trova riscontro in nessun altro Paese europeo (ad esempio la Germania, che rimpatria anche in Afghanistan), rischi di comportare una paralisi del meccanismo dei rimpatri, perché non ci sarebbero più Paesi da potersi considerare sicuri. Resta naturalmente indiscussa la prerogativa del magistrato di valutare nel caso concreto se quel Paese, sicuro in linea generale, lo sia nello specifico per il soggetto di cui poi si parla, spiegando, però, in maniera esaustiva e completa, caso per caso, quali siano le ragioni per cui, per un determinato individuo richiedente protezione internazionale, un determinato Paese non è ritenuto sicuro, passando, cioè, per usare le parole del presidente emerito della Consulta Mirabelli, da un'insicurezza tabellare ad un'insicurezza specifica in rapporto a un singolo individuo. Definendo un Paese insicuro in via generale, e non nel caso concreto, si rischia però di arrivare al paradosso di definire insicuri quasi la totalità dei Paesi del mondo, con la conseguenza di paralizzare il sistema delle procedure accelerate di frontiera, così come designato proprio dalla normativa europea. L'Italia si troverebbe, tra l'altro, nella situazione paradossale di dover rendere conto in sede europea della mancata tutela dei confini esterni dell'Unione. dell'Unione europea, infatti, afferma che non si può designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro soltanto per una parte di territorio. Solo in questo caso il giudice può, peraltro nel contesto della complessiva istruttoria, negare la qualificazione di Paese sicuro effettuata a livello nazionale, mentre è da escludersi che sulla base di indicazioni che attengono ad elementi diversi da quello della necessità che non ci siano deroghe relative a parti di territorio, il giudice possa disapplicare il decreto di individuazione dei Paesi sicuri che, come dicevo, attiene all'esercizio di una competenza espressamente riservata agli Stati membri proprio dalla direttiva del 2013. Ritengo che i giudici non possano disapplicare la legge siamo fiduciosi che in questa direzione andranno le determinazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, perché siamo certi di aver realizzato le procedure accelerate di frontiera esattamente così come previste dalla normativa europea. Tra l'altro, le procedure seguite dall'Italia anticipano di alcuni mesi, con l'approvazione del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, il nuovo regolamento UE 2024/1348

e prevederà criteri molto più diretti di qualificazione dei Paesi sicuri, legandoli al numero di domande di asilo accolte in tutta l'Unione europea. La necessità di individuare per legge i Paesi sicuri si inquadra nell'ambito del rafforzamento del sistema dei rimpatri, proprio per completare l'azione proficua che stiamo svolgendo per contrastare le partenze irregolari. Questo rafforzamento è un obiettivo richiesto dalla stessa Unione europea, come ha sottolineato anche la presidente von der Leyen in una lettera ai capi di Stato e di Governo, quando ha parlato di necessità di continuare a esplorare possibili strade da percorrere per quanto riguarda l'idea di sviluppare *hub* di rimpatrio al di fuori dell'Unione europea, evidenziando peraltro che, con l'avvio delle operazioni previste dal protocollo Italia-Albania, potremmo anche trarre lezioni da questa esperienza pratica. Albania, ieri tanto citato in quest'Aula, l'Italia si fa interprete come apripista del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. Sin dal momento della firma del protocollo fra Roma e Tirana, l'Europa guarda con interesse a questo accordo concluso tra l'Italia e l'Albania. A maggio 2024, 15 Stati membri dell'Unione europea, cioè più della metà considerato che sono in totale 27, hanno inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere maggiori sforzi nella gestione dell'immigrazione irregolare, in particolare attraverso accordi paritari e di lungo periodo con i Paesi di origine, sul modello di quello concluso con la Tunisia e l'Albania. L'attenzione riservata al progetto da 15 Paesi dell'Unione europea e dalla stessa Presidente della Commissione è la maggiore riprova del valore sperimentale e innovativo di un'iniziativa che si prefigge di contrastare l'immigrazione illegale senza incidere sulle garanzie e i diritti fondamentali delle persone, nella consapevolezza che ormai si va sempre più consolidando in Europa e che occorre affrontare la dimensione esterna delle migrazioni e la protezione delle frontiere, anche in collaborazione con gli altri Stati. Non me ne vogliate, ma mentre una parte

per il contenimento dell'immigrazione irregolare e il contrasto alla tratta di esseri umani. Per quanto riguarda le risorse investite (tanto citate) nei centri in Albania, lo stanziamento previsto, a seconda della variabilità del funzionamento delle strutture legata all'andamento dei flussi migratori, potrà certamente rivelarsi superiore ai costi effettivi. Però dobbiamo chiarire che questo milione (che poi sono 700) è riferito ai cinque anni, mentre nella comunicazione ho sempre sentito

tiene conto della collocazione geografica delle strutture. Va peraltro considerato che riguarda un impianto polifunzionale, un *unicum* che assolverà ad una quadruplice funzione: *hotspot* di sbarco, luogo di trattenimento e procedure accelerate, CPR e struttura carceraria. La somma stanziata corrisponde al 7,5 per cento delle spese connesse all'accoglienza dei migranti nel territorio nazionale nel 2023, che si è aggirata

si tratta, piuttosto, di un investimento che sul lungo periodo dovrà consentire di abbattere le spese di gestione e di prima accoglienza straordinaria. Quanto alle polemiche sui costi dei trasferimenti dei migranti nei centri in Albania con assetti navali pubblici, posso dire che si tratta di spese inferiori a quelle che sono state citate più volte, se si tiene conto che i numeri delle operazioni di analogo tipo nell'ultimo decennio evidenziano una media di centinaia di interventi l'anno, con punte di arrivi, in determinati periodi, che hanno gravato in maniera eccezionale sugli oneri a carico della finanza pubblica, nonché sul sistema dell'accoglienza. Come ha già avuto modo di evidenziare il ministro Piantedosi rispondendo ad alcune interrogazioni, si tratta di un fardello economico (che solo nel 2023 ammontava circa 2 miliardi di euro), oltre che gestionale, che il Governo in carica ha ereditato dalle epoche caratterizzate dall'assoluta mancanza di contrasto agli arrivi massicci e incontrollati. Il costo reale dell'impegno della nave Libra si è rivelato di 8.400 euro complessivi, al netto delle spese di ordinario esercizio quotidiano della nave; un costo giornaliero ampiamente inferiore a quello che veniva sostenuto nell'epoca della grande celebrazione di operazioni come Mare nostrum, che richiedevano oneri per 300.000 euro al giorno. È evidente che questa iniziativa ha anche una funzione deterrente, dimostrata dal fatto che nei primi nove mesi del 2024 i migranti arrivati irregolarmente in Italia in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. È ragionevole pensare che con l'entrata in funzione dei centri in Albania gli arrivi in Italia diminuiranno ulteriormente, con un conseguente contenimento complessivo dei costi. Anche le polemiche sul rispetto dei diritti dei migranti sono del tutto pretestuose, sia perché sono esclusi dal trasferimento nei centri in Albania donne, minori e soggetti fragili, per i quali resteranno naturalmente in piedi le regole previste dall'attuale normativa, che ne prevede l'accoglienza presso la rete del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI), sia perché il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli dei migranti, è tra i fondamenti dell'accordo siglato tra Roma e Tirana. Il fatto che nei predetti centri verranno espletate procedure di richiesta d'asilo, all'esito delle quali si stabilirà chi avrà il diritto di ottenere protezione internazionale e chi invece dovrà essere rimpatriato, è coerente con la normativa internazionale ed europea sul divieto di respingimento. Come ribadito dal presidente Meloni, sapevamo che avremmo incontrato numerosi ostacoli e un'opposizione molto più ampia, proveniente da vari ambienti che non sarebbero certamente stati d'accordo con questa iniziativa. tuttavia che non ci si debba fermare, mantenendo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ieri avete ovviamente sottolineato la parte che riguarda le corti d'appello. Sulla previsione introdotta alla Camera, che sposta dalle sezioni dei tribunali specializzati in materia di immigrazione alle corti d'appello in composizione monocratica la competenza sulla convalida del trattenimento disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, è utile ribadire che l'appello dei presidenti delle corti e dell'Associazione nazionale magistrati è stato frutto di una disattenzione, di una lettura poco attenta. Lo stesso presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, lo ha successivamente ammesso, parlando di confusione. Il ripristino dei ricorsi contro il respingimento delle domande d'asilo in corte d'appello, presente nella versione originaria del decreto flussi, è stato infatti soppresso con l'emendamento che trasferisce alle corti d'appello la competenza sulle convalide dei trattenimenti. L'intervento, quindi, alleggerisce gli uffici di secondo grado della prima materia, in modo da rendere sostenibile l'assegnazione alla seconda, evitando così il sovraccarico per le corti. Allo stesso tempo, viene innalzata ad un giudice superiore la cognizione rispetto ad una materia che tratta anche di diritti umani. diritti umani. Avete sottolineato la parte che riguarda i dispositivi elettronici. La norma che disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi e supporti elettronici o digitali in loro possesso, ovvero la loro ispezione, si ispira alla direttiva *2013**/**32**/**UE*. Essa consente agli Stati membri di prevedere disposizioni a livello nazionale volte a consentire alle autorità competenti di perquisire il richiedente ed i suoi effetti personali, nei quali rientrano anche e pacificamente i dispositivi o i supporti elettronici. La nuova norma introduce l'obbligo per lo straniero di collaborare nella ricostruzione della propria identità, fornendo informazioni su età, cittadinanza e Paesi di transito e consentendo, se necessario, l'accesso a dispositivi elettronici personali. Quest'obbligo è finalizzato a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il rischio che individui con falsa o incerta identità circolino sul territorio nazionale. L'ispezione L'ispezione autoritativa è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo per lo straniero rintracciato, in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro di attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento), o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, o minore straniero non accompagnato. L'ispezione così prevista è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche SIM e digitali in possesso dello straniero, nonché a documenti contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali, escludendo espressamente corrispondenza e comunicazioni personali. La procedura è rigorosamente circoscritta per rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione italiana. Sono consultabili solo dati rilevanti per l'identificazione e il percorso dello straniero. Inoltre, la norma prevede il controllo giudiziario successivo. I dati acquisiti senza convalida sono inutilizzabili. Lo straniero può assistere all'ispezione avendo accanto un mediatore culturale e un verbale dettagliato garantisce la trasparenza. Questa normativa è conforme alle leggi europee sul trattamento dei dati personali, stabilendo scopi, limiti e meccanismi di tutela. Francamente, è difficile giustificare, se non con un atteggiamento ostruzionistico e qualche volta strumentale, l'opposizione ad una norma che riveste grande importanza ai fini della salvaguardia della sicurezza dei cittadini, cui vogliamo dare priorità, assicurando sempre il bilanciamento con la tutela dei diritti di riservatezza dei migranti dei quali c'è la necessità di ricostruire l'identità. Abbiamo sollevato un tema che riguarda il ricongiungimento familiare, voluto da un emendamento proposto alla Camera, in 1a Commissione, dal collega Iezzi. L'articolo 12-*bis,* nel testo licenziato dalla 1a Commissione, impone la condizione di una residenza in Italia di almeno due anni per poter chiedere il ricongiungimento familiare. Da questa norma sono stati esentati gli stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno conseguente alla protezione internazionale. Con il diritto di ricongiungimento familiare senza condizioni si possono verificare e si sono verificate - situazioni abbastanza discutibili: lo straniero appena arrivato chiede il ricongiungimento con i suoi familiari, che, appena arrivati, a loro volta chiedono il ricongiungimento con altri familiari e così via, a catena. In sostanza, se c'è una ragione per fare entrare il primo, si determina una catena che consente di entrare in Italia

la parte che riguarda le sanzioni alle ONG. La norma relativa risponde all'esigenza di rafforzare il procedimento di erogazione della sanzione accessoria del fermo della nave, come oggi previsto, e di superarne alcune rigidità, come ad esempio la sua determinazione in misura fissa, questione recentemente sollevata per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale, rimettendo al prefetto l'applicazione e la determinazione della durata. In particolare, si restituisce organicità alla fase sanzionatoria della norma, con riguardo ai numerosi provvedimenti dell'autorità giudiziaria che ne hanno ripetutamente sottolineato l'inadeguatezza, sospendendo tutte le sanzioni accessorie, combinate dagli organi accertatori. Il testo, così come novellato, prevede ulteriori a beneficio degli eventuali trasgressori, sia in termini di riduzione della durata della sanzione accessoria, che viene definita in modo graduale all'interno di una forbice compresa tra un minimo e un massimo, sia riguardo allo snellimento della procedura e alle connesse garanzie procedimentali e alla tutela degli interessati, sia con riferimento all'autorità preposta all'adozione della sanzione amministrativa accessoria individuata nel prefetto. Infine, viene definita in modo più puntuale la disciplina della reiterazione degli illeciti commessi in violazione del novellato articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. Viene specificato che per reiterazione della violazione si intende una nuova violazione commessa

normativo si pone come il tassello essenziale di una strategia più ampia e articolata, che mira a dare alle istituzioni il controllo di un fenomeno epocale come quello delle migrazioni, finora lasciato in mano ai trafficanti e agli sfruttatori. Cosa vuole fare questo Governo? Vogliamo segnare il cambio di rotta rispetto a chi nei decenni si è disinteressato di ogni possibilità di regolamentazione, una visione ideologica che purtroppo ha prodotto solo insicurezza, emarginazione e sfruttamento. Il nostro obiettivo è chiaro: è costruire un sistema che consenta ingressi legali e sicuri, garantisca dignità, diritti e opportunità di integrazione a chi arriva e, allo stesso tempo, tuteli le nostre comunità dalla criminalità e dall'illegalità. è il senso del nostro impegno: governare le migrazioni in modo responsabile, promuovendo un modello sostenibile e soprattutto rispettoso dell'umanità delle persone, sia di chi arriva, sia soprattutto di chi accoglie. Solo attraverso regole chiare, solo attraverso azioni concrete, infatti, possiamo realmente coniugare sicurezza, legalità e solidarietà, costruendo un meccanismo di regole grazie al quale le immigrazioni potranno rappresentare davvero un'opportunità di crescita per chi arriva in Italia e per la nostra comunità nazionale. Chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi per tutto questo tempo - forse ne ho preso troppo - ha sentito il mio accento e capisce che vengo dal profondo Sud, quindi sinceramente da donna orgogliosamente meridionale, anzi orgogliosamente terrona, per il mio attaccamento alla terra, non accetto nessuna accusa rispetto alla crudeltà e a qualsiasi forma di razzismo: noi siamo emigrati per lavorare, siamo emigrati per curarci, siamo emigrati per studiare, sappiamo esattamente cosa significa lasciare la propria terra. È altrettanto vero che ci possiamo spostare dalla nostra terra, ma quella terra non la può togliere nessuno da dentro di noi. Dobbiamo comunque farlo con la consapevolezza che le regole sui diritti non si possono mettere in discussione. Auspico, quindi, ovviamente sapendo già quale sarà l'esito del voto, che ci sia la volontà

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge

Non possiamo non rilevare e stigmatizzare la singolarità dell'intervento che abbiamo ascoltato in questo momento da parte della rappresentante del Governo, una doppia singolarità dal punto di vista strettamente formale e nel merito, su cui poi per noi interverrà il presidente Renzi. Non può non colpire il fatto che la rappresentante del Governo (che noi abbiamo ascoltato con grande attenzione,

come se fosse la relatrice di questo provvedimento e a questo punto coglie bene l'*iter* di tutta questa vicenda, perché va ricordato che questo provvedimento è arrivato in Aula senza che il relatore abbia avuto il mandato da parte della Commissione, la quale è stata aperta e chiusa nel giro di un'ora, senza neppure avere la possibilità di affrontare l'esame degli emendamenti proposti dalle opposizioni. Mi pare quindi di tutta evidenza che il Governo è stato costretto a tornare, almeno dal punto di vista dell'impostazione, sui propri passi, venendo in questa sede per tentare di giustificarsi rispetto ad una prassi che ha, per l'ennesima volta, strozzato la libertà di quest'Assemblea di entrare nel merito dei provvedimenti. La seconda cosa piuttosto singolare che colpisce è che la rappresentante del Governo in questa sede ha fatto - lessicalmente - lo stesso intervento che ha fatto alla Camera

che sta dall'altra parte. *(Applausi)*. Io vorrei darle una comunicazione di servizio: ieri sono intervenuti diversi senatori. Avrebbe almeno potuto fare lo sforzo di farsi passare, se non direttamente di appuntarsi, i nomi di coloro i quali ieri sono intervenuti, come il senatore Scalfarotto, il senatore Delrio, la senatrice Musolino. Insomma, tanti hanno dato il proprio contributo; si è, invece, evocato (magari per far tornare alcuni equilibri all'interno della maggioranza, un po' scricchiolanti di questi tempi) l'onorevole Iezzi, come è noto non appartenente a questo ramo del Parlamento. quindi introdotto una innovazione ulteriore: il Governo impedisce all'Assemblea di esprimersi, strozza il dibattito con la fiducia, viene qui con un compitino preconfezionato, che manda qualche pizzino all'interno della maggioranza, e finisce con un fervorino. Grazie dell'innovazione.

Signora Presidente, onorevoli colleghi del Senato, signor Ministro, signora Sottosegretaria, non posso che riprendere ciò che ha detto il collega Enrico Borghi. Sottosegretaria, io ho...

Senatore Renzi! Inizio con i richiami. Non siamo allo stadio e non state dando una grande prova di educazione davanti ai ragazzi del liceo in visita. *(Applausi)*. Per cortesia, senatore Renzi, lei ha la possibilità di parlare in dichiarazione di voto.

non mi consentirei mai di accusarla di razzismo o di cattiveria; però, se il Governo deve intervenire in risposta a un dibattito, si chiede che intervenga in risposta al dibattito che c'è stato qui al Senato. È una questione di rispetto per le nostre prerogative, per tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che sono intervenuti ieri. Siamo nuovamente chiamati a pronunciarci sul tema che più di ogni altro è alimentato dal furore ideologico nel nostro Paese: l'immigrazione. Siamo all'ennesimo provvedimento di questo Governo sul tema dell'immigrazione: il decreto Cutro, il decreto Italia-Albania, ora il decreto flussi. Sono otto i decreti che in due anni, dall'inizio della legislatura, hanno avuto per tema principale l'immigrazione e ogni volta ricorrete alla decretazione d'urgenza, perché non riuscite ad affrontare il tema dell'immigrazione in una prospettiva che non sia di carattere emergenziale. In questo provvedimento confluiscono due macrotemi: quello della lista dei Paesi sicuri, che viene emendato dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, e quello del decreto flussi. Sul primo aspetto, torno a ribadire che la sentenza dei giudici europei non dice nulla di eclatante, se non che la lista dei Paesi sicuri è di competenza degli Stati membri, che va fatta tenendo conto che le condizioni di sicurezza all'interno di un Paese possono variare nello spazio e nel tempo… *(Brusìo)*. PRESIDENTE. Senatore Lombardo, le chiedo per cortesia di fermarsi. Allora, facciamo così: se non c'è silenzio in Aula, io fermo i senatori ogni volta. Come dicevo, il concetto di sicurezza varia nello spazio territoriale, nel tempo e nelle condizioni sociali del richiedente. La Sottosegretaria ha detto che adesso passiamo da un decreto ministeriale a una norma di legge. La Sottosegretaria sa benissimo che il diritto nazionale, anche qualora abbia una legge, se in contrarietà col diritto europeo, può essere disapplicato dai giudici nazionali. Non è la forma, non è il decreto ministeriale o la norma, ma è il contenuto. Se volete garantire la certezza del diritto rispetto alla disapplicazione dei giudici nazionali per contrasto al diritto dell'Unione europea, non basta questo nuovo intervento normativo. Serve che abbiate la forza politica di portare la normativa a livello europeo, con una lista europea di Paesi sicuri che garantisca uniforme applicazione e interpretazione del diritto. Il secondo elemento di cui si compone questo decreto riguarda i flussi migratori. Qui io non penso che voi siate razzisti, non penso che siate cattivi. Penso che l'intervento normativo sia completamente fuori fuoco rispetto a quello di cui avremmo bisogno oggi in Italia. L'attenzione politica si concentra sugli sbarchi, mentre dovrebbe concentrarsi sulle partenze e sulle modalità di accesso. Il sistema legale di ingresso dei migranti in Italia, basato sulle quote dei flussi e sul *click day*, non funziona. Non funziona, perché è incivile stabilire che il destino di un uomo dipende da un *click*; non funziona perché quel *click* è in mano talvolta alle organizzazioni criminali, come dimostrano talune inchieste giudiziarie che sono state citate dalla Sottosegretaria; non funziona perché si limita a regolarizzare chi è già in Italia e non regola i flussi dei migranti che vogliono arrivare nel nostro Paese. La possibilità di far entrare 10.000 persone per l'assistenza domiciliare - chiamiamola con il suo vero nome - non si chiama sperimentazione, si chiama sanatoria. Si chiama sanatoria di badanti stranieri che già oggi sono nel nostro territorio e vivono nelle nostre case, ma non è procedendo di sanatoria in sanatoria che contrasteremo l'immigrazione clandestina. C'è un modo per contrastare l'immigrazione irregolare nel nostro Paese. Qual è il modo più efficace per contrastare l'immigrazione irregolare nel nostro Paese? Favorire canali di migrazione legale, regolare e sicura *(Applausi)*.

per favorire la formazione a distanza nei Paesi di origine. Il quarto punto si chiama difendere i corridoi umanitari, che devono essere riservati ai richiedenti asilo e protezione internazionale, perché sono coloro che scappano da persecuzioni e da guerre ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il quinto è contrastare l'immigrazione irregolare con l'espulsione e l'obbligo di rimpatrio per coloro che arrivano nel nostro territorio violando la legge nazionale. Conosco l'obiezione: perché pensare ai lavoratori migranti stranieri e non mettere prima gli italiani? La risposta è semplice, è molto semplice: un esercito di lavoratori irregolari stranieri abbassa le condizioni di lavoro per tutti, inclusi gli italiani. Finché esisterà un esercito di lavoratori in nero, migranti sottopagati che accettano di lavorare a basso costo, senza sicurezza e senza tutele, la concorrenza nel mercato del lavoro sarà sempre al ribasso e chi ci perderà saranno sempre le imprese oneste, che rispettano le leggi e i lavoratori, siano essi italiani o stranieri. Se portiamo alla luce e alla legalità l'economia sommersa, che rappresenta per fatturato la più grande industria italiana, avremo riportato condizioni più eque di lavoro per tutti, stranieri ed italiani. È per questo che avevamo presentato, a firma mia e del senatore Carlo Calenda, un emendamento all'articolo 1 che intendeva introdurre nel nostro ordinamento giuridico un meccanismo permanente di regolarizzazione degli stranieri, ovvero il permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale, quando un lavoratore straniero, ancorché presente irregolarmente nel nostro territorio, sottoscrive un contratto di lavoro subordinato non inferiore a un anno. Un intervento sistemico per far emergere il lavoro nero e contrastare il fenomeno del caporalato, dello sfruttamento e dell'intermediazione illecita di manodopera. Questa visione manca totalmente in questo provvedimento. Ci sono cose positive, come la semplificazione del *click day*, ma non c'è il coraggio di abolirlo. Ci sono poi storture che rischiano di peggiorare. Lo spostamento della competenza sul trattenimento dei migranti alle corti di appello rischia di portare le corti al collasso, con un aumento dei carichi di lavoro dei magistrati fino al 30 per cento, secondo le simulazioni dell'ufficio studi del La parte in cui voi modificate il sistema di accoglienza, avendo in mente l'ipotesi che fa più clamore, quella del soccorso in mare, si dimentica di chi viene da terra. L'ipotesi di vincolare la risposta delle prefetture alle rotte marittime, dando priorità di accoglienza a chi viene gestito dagli *hotspot* del Ministero dell'interno, vi sta facendo perdere di vista la necessità di rafforzare la presa in carico della rotta balcanica, dove transitano silenziosamente profughi afgani e siriani. Ascoltate gli amministratori di quei territori che trovate lungo la A4; ascoltate l'appello che hanno mandato a tutti i parlamentari. Così state creando ulteriori disparità nel sistema di accoglienza. Arrivo a concludere, signora Presidente, e la ringrazio del minuto in più che mi ha dato. Una gestione politica dei flussi migratori, oltre la dittatura dell'emergenza, oltre la logica securitaria che vede nell'immigrazione solo una minaccia, significa investire nella formazione e nell'inclusione dei migranti e promuovere una convivenza civile, basata sul rispetto della legge e soprattutto sul rispetto della dignità degli uomini, a prescindere dalla nazionalità da cui provengono. Per questi motivi, annuncio il voto contrario di Azione al provvedimento in esame. Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, se il Parlamento nelle democrazie liberali ha un senso, è perché qualcuno vi parla e qualcuno ascolta. Noi oggi abbiamo ascoltato una controrelazione della Sottosegretaria e l'abbiamo fatto in silenzio, a differenza dei banchi della maggioranza. Non l'abbiamo condivisa, facendo un richiamo al Regolamento del tutto legittimo e rispettabile, e abbiamo evidenziato i nostri dubbi su come si è concepito il dibattito parlamentare in quest'Aula. A fronte di questo, le provocazioni, le minacce, il roteare le mani, come ha fatto un parlamentare della maggioranza mentre parlava un parlamentare dell'opposizione, "fate i bravi, ne riparliamo dopo", ma è un atteggiamento che svilisce la funzione per la quale tutte e tutti siamo qui che è quella di votare delle leggi sulla base di un ascolto reciproco e di una valutazione nel merito che noi abbiamo fatto ascoltando il Governo, e che la maggioranza, almeno in alcuni suoi elementi, ha inteso non fare. Per questo, Presidente, mi sono accalorato nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza: perché compito della Presidenza è quello di garantire alle opposizioni il diritto di portare la propria voce, a maggior ragione quando questo avviene in una cornice istituzionale quale quella che il presidente Enrico Borghi ha ricordato poc'anzi, ossia di sostanziale impedimento al lavoro in Commissione. Vengo all'intervento, fatta questa doverosa premessa che un servitore delle istituzioni ha il dovere di fare e che sono certo troverà accoglimento in larga parte della maggioranza, colleghi perbene e persone serie che condividono - anche se non lo possono dire - quello che ho appena detto. Vengo al testo che mi ero immaginato, anche alla luce di ciò che ha detto la sottosegretaria Ferro. Diceva Niccolò Machiavelli, che era un segretario fiorentino di quelli seri, che governare è far credere, e voi in questo siete bravissimi, signori del Governo. Voi fate credere che l'immigrazione irregolare sia il problema di questo Paese. Voi oggi siete in una fase di scontro con i sindacati; bene, ascoltate gli imprenditori che vi dicono che abbiamo un problema di immigrazione, sì, ma abbiamo un problema di scarsa immigrazione regolare. E, nel far credere che tutto il dramma di questo Paese sia l'immigrazione irregolare, riuscite con abilità straordinaria - vi faccio i complimenti - a cancellare le notizie. Oggi cito «Il Giornale»

e come nel mese di novembre siano aumentate del 4,6 per cento. Ma il tema delle bollette non esiste, perché c'è l'immigrazione irregolare. Le liste d'attesa, su cui avete fatto un decreto inutile a giugno, sono sempre più un problema. Ma voi non lo fate considerare, perché il problema è l'immigrazione irregolare. I vostri figli non trovano casa a Milano perché gli affitti sono troppo alti? Non è un problema, tanto basta metterci una bella passata di immigrazione irregolare e governare facendo credere che questo sia l'unico problema. Questa narrazione è efficace. Vi racconto un fatto. Signora Presidente, due giorni fa partecipavo a una trasmissione televisiva su Rete 4, non propriamente una trasmissione che potremmo definire di sinistra. Mi fermo a parlare con il pubblico in studio, al termine della trasmissione, e mi metto a discutere. Quasi tutti hanno idee diverse dalle nostre, ma ci mettiamo a parlare, è bello, è sempre piacevole. Al che una signora mi dice, a telecamere spente: «Tanto tu devi stare zitto, perché gli immigrati irregolari in Italia li hai fatti venire tu, tutti nel 2015». 2015». Perché la narrazione, efficacissima, è stata che Renzi ha aperto le porte agli immigrati e nel 2015 siamo stati invasi. Allora guardiamo i numeri, per vedere se è vero. Immigrazione irregolare, sbarchi nel 2015 in Italia, Governo Renzi: 153.000. Tantini, sì. Immigrazione irregolare, sbarchi, Governo Meloni, 2023: 158.000. Cioè la Meloni ha avuto, nell'unico anno solare pieno di Governo (per il momento), più sbarchi di quanti ne ho avuti io nell'unico anno pieno di Governo. Però questi numeri non passano fuori, perché la narrazione è: «Noi combattiamo l'immigrazione irregolare!». Solo che, a un certo punto, c'è un problema da porsi: come si fa a combatterla? Ecco che qui arrivano il talento, il genio, l'innovazione, la fantasia: apriamo un centro migranti in Albania. Il centro migranti in Albania è una delle più grandi buffonate che si potessero immaginare in questa storia parlamentare. *(Applausi)*. E non per questioni regolamentari e giuridiche, su cui brevemente arriverò tra poco, ma per questioni numeriche. ma per questioni numeriche. Ci siamo permessi di correggere, venendo in aiuto alla sottosegretaria Ferro: la cifra che noi contestiamo è un miliardo e giustamente lei subito lo ha evidenziato, dicendo che secondo lei sono meno (vedremo, faremo i conti a consuntivo). Ma che siano 700 milioni, come dice la Ferro, o che sia un miliardo, come diciamo noi, sono tanti soldi che vengono sottratti al bilancio pluriennale dello Stato e messi a disposizione di un centro migranti in Albania, che oggi la Sottosegretaria ha voluto definire, con un'espressione che io condivido, «centro polifunzionale». (L'abbiamo ascoltata). È un centro talmente polifunzionale - signora Sottosegretaria, lo dico a lei per il tramite della Presidente - che oggi svolge la funzione di canile per i cani randagi, che stanno occupando il centro polifunzionale per migranti costato un miliardo di euro del contribuente. *(Applausi)*. Tale centro oggi non sta dando riparo a nessun migrante, ma a tanti cani randagi albanesi, la cui sorte ci sta a cuore. Ma a me - prenderò le accuse degli animalisti - la sorte dei cani randagi albanesi sta meno a cuore della sorte degli operai italiani che devono, con le loro tasse, pagare la vostra propaganda e la vostra ideologia. allora vengo ai temi di merito. La vostra narrazione si scontra con la realtà, perché non state risolvendo il problema dell'immigrazione, ma state sprecando poliziotti e carabinieri che servirebbero nelle nostre stazioni, nelle nostre periferie, nelle nostre strade, i quali sono costretti a stare nei quattro stelle o nei cinque stelle albanesi albanesi ad attendere che il tempo passi. Avete instaurato l'unico sistema di pendolari che funziona in Italia *(Applausi)*, perché, da quando c'è Salvini non funziona e non arriva in orario più un treno, non è in orario più un Frecciarossa, ma come è puntuale il traghetto tra la Puglia e l'Albania, che porta il migrante e lo riporta indietro alla luce delle sentenze! Non c'è niente di così ordinato e regolare in Italia, nel trasporto pubblico, quanto la nostra struttura della Marina che va a prendere i migranti e ne riporta sette per volta. A fronte di questo, signora Presidente, voi avete sottovalutato i veri problemi che ci sono. Ne cito tre e concludo. Avendo scelto di aprire uno scontro con la magistratura, fatevelo dire da un esperto: con la magistratura ci si può scontrare e, in alcuni casi, ci si deve scontrare, scontrare, ma con la magistratura, se si è dalla parte di quelli giudicati responsabili o colpevoli, ci si scontra con i ricorsi in aula, non andando in Parlamento e facendo le leggi contro di essa. *(Applausi)*. Io, quando sono stato indagato ingiustamente, non è che sono venuto in Parlamento a dire fatemi una leggina perché ce l'ho con i magistrati, sono andato in aula e ho presentato una denuncia penale contro i magistrati che ritenevo avessero violato le leggi. Così si fa, non è che si patteggia e poi si viene in Aula a cercare di cambiare le cose. Se volete uno scontro con la magistratura, rispettate la separazione dei poteri, andate in aula e fate provare lì cosa significa avere realmente a cuore le istituzioni. *(Applausi)*. Voi no, avete scelto un *ping-pong* con la magistratura perché vi serve. serve. Se non siete perseguitati infatti vi dimostrate incapaci, cioè inidonei a risolvere il problema dell'immigrazione. Ecco perché vi serve lo scontro con la magistratura. Serve a voi più che alla magistratura. I tre punti e concludo. Il primo: c'è un tema di sicurezza, signora Presidente, in questo Paese e lo deve capire anche la sinistra radicale; in alcuni casi, alcuni suoi esponenti, appena ritornati dall'occupazione abusiva delle case, hanno scelto di giustificare la violenza al Corvetto. La questione della sicurezza non si può lasciare alla destra, ma riguarda l'intero arco costituzionale. Se noi non siamo duri con il crimine e con le cause del crimine, non saremo mai capaci di essere alternativi a una visione ideologica come quella che ha il centrodestra. Il professor Billari, rettore della «Bocconi», demografo tra i principali al mondo, ha citato numeri che vorrei ci facessero riflettere; il 67,5 per cento degli studenti stranieri che frequenta le nostre scuole è nato in Italia;

o rischiamo la stessa identica situazione che aveva la Francia dieci anni fa; ero al Governo e ricordo le *banlieue* in fiamme, gli attentati terroristici al Bataclan e alla sede O interveniamo con la coesione, l'educazione, le risorse in cultura e in sicurezza, tenendo insieme la legalità e l'investimento educativo, o perdiamo una generazione *(Applausi)*, che non è quella dei poveri cristi che stanno sbarcando, ma quella dei figli delle seconde generazioni. Ultimo punto:

In Siria c'è un popolo disintegrato da anni, lustri di guerra. C'erano due milioni di cristiani nella culla del cristianesimo. San Paolo cade da cavallo sulla strada verso Damasco, è la Siria la culla della cristianità, dove vi erano due milioni di cristiani, adesso ce ne sono 500.000. Sono stati resi martiri dalla follia e non è che quelli che sono appoggiati dalla Russia sono cattivi e gli altri sono buoni. buoni. Quelli contro cui stanno combattendo i russi e gli iraniani sono i brigatisti tagliagole del Daesh, dello Stato islamico, dell'Isis. Bisogna avere il coraggio di dire che non si può essere superficiali in politica estera. A fronte di questo io sento, da italiano, da uomo che crede nelle radici cristiane di questo Paese, il dolore per il popolo siriano; 500.000 cristiani ancora massacrati e noi abbiamo un Ministro che, come unica cosa che sa dire di fronte al disastro siriano, è che siamo preoccupati per il collasso migratorio. Amici e colleghi, Amici e colleghi, amici e compagni di qua, o noi abbiamo il coraggio di ricordarci che di fronte a ciò che sta avvenendo nel mondo, non c'è bisogno soltanto di far credere, ma anche di fare politica, possibilmente anche di fare un po' di politica estera, oppure voi continuerete a prendere occasioni come queste e rendere sostanzialmente uno *spot* ideologico e uno spreco di risorse quella che poteva essere una grande iniziativa *bipartisan*. Ritornate in voi e recuperate la dignità della politica.

Signora Presidente, spiace che in quest'Aula si sia assistito oggi a questa esagitazione proprio su un provvedimento che interessa moltissimo gli italiani. Mi piacerebbe poi dire al senatore Renzi, che parla di far credere e ha citato i numeri del Governo Meloni, che nel 2024 il Governo Meloni ha fatto

Signora Presidente, onorevoli colleghi, sin dal suo insediamento il Governo Meloni, come da promesse fatte agli italiani (che noi siamo soliti mantenere), ha posto tra i suoi obiettivi primari il contrasto all'immigrazione irregolare, una priorità di tutta la maggioranza di centrodestra che sostiene questo Esecutivo, perché non è più oggettivamente pensabile che l'Italia da sola possa fronteggiare questo drammatico fenomeno che alimenta il deplorevole *business* dei trafficanti di esseri umani, con tutto il bagaglio di disagio che ne deriva a cittadini e immigrati stessi, che spesso finiscono a fare una vita peggiore di quella dalla quale sono scappati. Non ci si può nascondere, non si può mentire ad una opinione pubblica esasperata. Dobbiamo avere il coraggio di dire che la gestione dei flussi illegali è nelle mani delle organizzazioni criminali e che un Governo ha il dovere di affrontare questo tema senza pregiudizi e di fermare quei barchini che troppo spesso si trasformano in trappole mortali, lasciando nel Mediterraneo, che diventa il loro cimitero, corpi senza vita e purtroppo senza nome, di chi si è affidato o è stato costretto ad affidarsi alla parte sbagliata. *Ergo*, come si combatte l'immigrazione illegale? Paradossalmente lo hanno detto anche i colleghi che mi hanno anticipato, però lo hanno messo in negativo, mentre la soluzione messa in campo dal Governo Meloni assolutamente positiva. Lo si fa solo con flussi migratori regolari e legali. Così si combatte l'immigrazione. Possiamo farlo sovrapponendo l'ingresso dei lavoratori extracomunitari alle ingenti necessità di manodopera richiesta dal tessuto produttivo imprenditoriale italiano. È un nuovo approccio, l'unico forse possibile: pensare all'immigrazione prevedendo la possibilità di individuare nei Paesi d'origine quella manodopera da formare nei luoghi di provenienza, per procedere solo in seguito all'ingresso nel nostro territorio. La rotta dei trafficanti di morte punta all'Italia; la rotta del Governo del Governo Meloni punta alla legalità e a regole certe per salvare vite umane e la civile convivenza nel nostro Paese. Non solo salvarle da viaggi a rischio, in condizioni disumane e inaccettabili, soprattutto per donne e bambini, ma per tutelare chi arriva e non lasciarli nelle mani della criminalità, che continuerà a sfruttarli, magari a causa di debiti contratti per il viaggio. organizzazioni criminali costringeranno le donne a vendere i propri corpi, trasformeranno in schiavi gli uomini da mandare nei campi, renderanno prigionieri della droga giovani che faranno i galoppini per smerciare sostanze stupefacenti. L'illegalità genera insicurezza e l'insicurezza porta degrado. Noi non ci arrendiamo a questo come dimostra l'approccio del Governo Meloni anche con il piano Mattei, che, oltre ad un approccio non predatorio, bensì formativo e di scambio di conoscenze con i Paesi del continente africano, ha portato il nostro Paese ad approvare relazioni bilaterali con i territori di partenza, senza dimenticare i protocolli per il centro migranti in Albania, momentaneamente (solo momentaneamente, senatore Renzi) contrastato da qualche giudice che dimentica di dover giudicare in nome del popolo italiano con obiettività, senza pregiudizio politico, e poi anche con Paesi come la Tunisia, l'Egitto, l'Albania e la Libia. Oggi attendiamo la sentenza, se non verrà appositamente rimandata. Tutto questo è frutto di un lavoro serio, preso ad esempio anche da altri Stati europei, come Germania e Inghilterra; altro che invenzione, altro che approccio disumano, altro che negatività, altro che follia. È un approccio nuovo, giusto, seguito da altri Paesi, che non porta a girarsi dall'altra parte lasciando soli gli uomini. Regole certe per la disciplina d'ingresso nel nostro Paese, come previste dal decreto-legge in esame, non erano più rinviabili. Con questo provvedimento introduciamo misure volte a semplificare e regolare i flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche e prevedendo l'eliminazione del silenzio assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Interveniamo con una corposa semplificazione, perché purtroppo alcune volte è nelle pieghe (e, se volete, nelle piaghe) della burocrazia che prolifica il malaffare. Incrementare le quote di ingresso per il lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, dando priorità a determinate categorie, è doveroso. Prima del Governo Meloni i decreti flussi su base triennale non erano approvati *ex ante*, ma *ex post*. Ciò vuol dire che prima si facevano entrare i cittadini extracomunitari e poi si procedeva con l'individuazione dei numeri da approvare con specifico decreto. Non c'era programmazione, ma un semplice visto, una presa d'atto di quanto già accaduto. Decidere prima, invece, porta ad una forma di protezione per i lavoratori stranieri e ad una sicura tutela contro i fenomeni di sfruttamento. Allo stesso tempo, siamo convinti che serva la repressione per fermare condotte criminose. Per questo estendiamo le pene per i reati di tratta e sfruttamento. Per operare, per intervenire servono risorse. Ecco perché si incrementa il fondo per le emergenze nazionali di cinque milioni per l'anno 2024 (comma 2) e si destinano 35 milioni per l'anno 2024 alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie. È doveroso stabilire regole certe anche per le imbarcazioni. In particolare, attraverso l'articolo 11 viene modificata la durata del fermo amministrativo della nave, applicato qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dall'autorità competente o non si uniformino alle loro indicazioni, stabilendo che venga disposto il fermo per un minimo di dieci fino ad un massimo di

Si prevede, infine, che, in caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro, nell'ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinino il mancato assolvimento da parte del richiedente dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare. Questo significa entrare nel merito delle cose, cari colleghi. L'articolo 15 assegna alla commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Non possiamo, infatti, negare l'evidenza dei fatti, come fanno spesso le opposizioni e lo abbiamo appena sentito. Moltissime persone straniere che vengono in Italia delinquono. Negarlo significa tradire le vittime di rapine, violenze e abusi da parte dei cittadini extracomunitari. Negarlo significa tradire il il nostro mandato di tutelare i cittadini italiani. La stucchevole polemica sui numeri degli autori di stupri, come elencati con puntualità e precisione da autorevoli Ministri di questo Governo, lascia basiti: o non si comprendono i numeri e lo stato d'animo di chi subisce violenza o si vuole raccogliere un tornaconto elettorale che proprio non si capisce da dove o da cosa possa derivare. Difendere chi commette un reato, infatti, significa tutelare indirettamente le organizzazioni criminali che illegalmente hanno portato in Italia chi ha scelto la strada della delinquenza e non quella dell'accoglienza dell'accoglienza e dell'inclusione. Sulla disciplina dei programmi di rimpatrio forzato si attribuiscono specifiche competenze alle corti d'appello per la convalida del provvedimento sul trattenimento dei richiedenti asilo, asilo, tenendo conto della provenienza dello straniero da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione. L'opposizione che fa le barricate perché si è attribuita ad un giudice di rango superiore la possibilità di decidere su un tema così delicato fa sorridere. Ringrazio chi ha ricordato, sbagliando, che questo provvedimento è contrario ai principi dell'Unione europea. Lo ringrazio, perché ci permette di fare una piccola lezione di diritto in queste aule ai disfattisti di professione. È uno Stato che ha il diritto e il dovere di elencare i territori sicuri o no. Accogliere un essere umano, colleghi, significa prendersene cura. Accoglienza significa inclusione ed inclusione significa integrare una persona in una comunità, garantirle gli stessi diritti, ma, allo stesso tempo, attendersi anche il rispetto dei doveri. Signor Presidente, concludo dicendo che il Governo Meloni sta lavorando in questa direzione. Una via nuova, ma soprattutto giusta, che allo stesso tempo difenda

sono stato corretto dal Governo: è l'ottavo provvedimento specifico in cui si affronta la questione immigrazione, ma diventa il diciassettesimo, se si considerano anche quelli in cui la vicenda

complessivamente abbiamo affrontato la questione immigrazione 17 volte, significa che in quest'Aula ce ne occupiamo una volta ogni mese e mezzo. È davvero molto indicativo il numero che sto dicendo:

Non lo dico io, ma lo dicono i dati Istat, che sono indiscutibili. Tanto per dirne una, vogliamo parlare del numero degli omicidi che ci sono stati nel nostro Paese?

746 nel 2000, 601 nel 2005, 526 nel 2010, 469 nel 2015

Quindi, non era semplicemente un problema di guerra di mafia. Il problema penso che sia inverso, ossia l'idea, che subiamo da molti anni a questa parte

anche le forze dell'opposizione e si scontra con i dati della realtà. Esattamente come dicevo poco fa, anche sui numeri dell'immigrazione bisogna dire la verità e fare chiarezza: non è vero che stiamo subendo un'invasione. Davvero si può parlare di invasione, se parliamo di poco più di 100.000 persone a fronte di 60 milioni di abitanti? Ma lo sapete quali sono i numeri che riguardano, invece, altri Paesi del mondo che - quelli sì - hanno avuto a che fare, anche perché sono confinanti, con fenomeni migratori in quel caso davvero clamorosi e davvero giganteschi? Peraltro, parliamo, come sapete, di un Paese in cui vengono rimpatriati 4.000 migranti all'anno. Penso che sarebbe opportuno - ma di questo non parliamo mai, perché evidentemente non è funzionale alla narrazione che viene fatta in quest'Aula - che si parlasse della difesa dei confini anche da un altro punto di vista. Per esempio, mi piacerebbe molto che parlassimo della difesa dei confini dal punto di vista delle decine di migliaia di giovani italiani che tutti gli anni dall'Italia se ne vanno. *(Applausi)*. Vogliamo citare i numeri anche su questo? Nel 2022, 150.000 italiani sono andati via dal nostro Paese. La verità è che il nostro è ancora un Paese di emigranti e di questo dovreste rendervi conto, perché purtroppo le giovani generazioni non sono tutelate come dovrebbero. Sappiamo, anche in questo caso, che parliamo di una emigrazione che non è nemmeno più quella con la valigia di cartone, ma coinvolge giovani laureati, giovani specializzati che sono costretti ad abbandonare il nostro Paese. Ma Ma di questo non parliamo, perché parliamo invece, per l'appunto, della invasione dei migranti, in una narrazione farlocca e fasulla che evidentemente è funzionale a costruire un'operazione di propaganda. E anche in questo decreto non si fa altro che insistere su questo tipo di argomento. Naturalmente, avete preso di mira - perché ne siete davvero ossessionati - un vostro nemico giurato, che sono le ONG, ma non è una novità. Alle ONG, che io invece voglio ancora una volta in quest'Aula pubblicamente ringraziare per il lavoro che fanno *(Applausi)*, voi volete vietare di utilizzare aeromobili per cercare di trovare le barche che stanno affondando. rivolgo al Governo: mi viene davvero il dubbio che abbiate paura di un'altra cosa. Signor Presidente, durante le audizioni alla Camera, la portavoce di Sea Watch, che è una ONG che tutti conosciamo, ha mostrato un video - devo dire - abbastanza drammatico, nel quale si vede con chiarezza che sulle motovedette che lo Stato italiano ha regalato ai libici,

su barche che voi avete dato alla Guardia costiera libica? Possibile che questa circostanza non intercetti la nostra coscienza e non parli di un problema grande e gigantesco? È possibile che dinanzi a questo si risponda vietando l'utilizzo di aeromobili e quindi in qualche modo impedendo che si possano vedere le ingiustizie e le torture che vengono perpetrate nei confronti dei migranti? A me pare molto indicativo quello che sta accadendo. Esattamente come mi sembra molto indicativa questa norma, che pure è contenuta all'interno del decreto, che prevede che debbano essere secretati i contratti per la fornitura di materiale a Paesi terzi, come la Libia per le motovedette o come l'Albania, perché deve rimanere tutto segreto. Anche a

aggiungere altre considerazioni che pure meriterebbero un approfondimento. Naturalmente prima fra tutte è quella sul fallimentare progetto dell'Albania, di cui spesso si è parlato, nascosto da elementi di poca chiarezza: un progetto o un provvedimento - non so nemmeno bene come definirlo - che, oltre a essere un vero e proprio abominio giuridico, almeno dal mio punto di vista, rischia di diventare anche uno dei più grandi sprechi di denaro pubblico della storia recente e passata. Buttiamo 700 milioni in Albania nello stesso momento in cui, nella legge di bilancio, investiamo per la scuola un miliardo. Ma possibile, davvero, che si possa dedicare a una cosa grande, gigantesca come l'istruzione pubblica, uno dei grandi temi di questo Paese, o alla sanità pubblica così poca considerazione e che invece dedichiamo tutto il tempo, tutti i soldi, tutte le risorse alla costruzione del nemico immaginario e del fantasma dell'immigrazione? Ecco, a me pare che su questo davvero occorra fare una grande operazione di verità. Noi non stiamo subendo un'invasione. Dovremmo avere il coraggio e la forza di ribaltare radicalmente il punto di vista. Io lo dico oggi a voi, ma non ho smesso di dirlo anche nel corso degli anni precedenti, anche quando governavano altri: noi dovremmo provare ad affrontare la questione dell'immigrazione con un altro sguardo, immaginandola come una risorsa, come una opportunità,

abrogare una volta per tutte quello che resta della cosiddetta legge Bossi-Fini, la legge che più di tutte le altre ci ha messo nella condizione negativa nella quale viviamo.

Intanto voglio dire che Forza Italia ritiene validissimo il provvedimento che è arrivato a noi, certo, con tempi un po' ristretti, per il famoso monocameralismo di fatto, tema che prima o poi dovremo affrontare. Tuttavia, alla Camera dei deputati - come capita a noi, al Senato, su altri provvedimenti - hanno avuto modo di fare un lavoro approfondito. Hanno sentito tutti, perfino Sea Watch, che è quella ONG che - secondo me - collabora a un'attività inopportuna e di incoraggiamento sostanziale dei trafficanti di persone. È stata sentita - e questa è stata una scelta più virtuosa la Guardia costiera, che con 11.000 donne e uomini dà un contributo fondamentale alla salvezza di vite umane e al contrasto all'attività dei trafficanti. Voglio quindi cogliere questa occasione per elogiare e ringraziare, una volta di più, la Guardia costiera. Vorrei che anche le ONG collaborassero di più, perché resta il fatto che molte ONG operano come fattori di attrazione; collaborano con i trafficanti di persone; hanno traffici telefonici e comunicativi che sono stati accertati e dimostrati; svolgono un'azione di concorso, morale e materiale con chi lucra sulla disperazione degli immigrati. Questa è la realtà. *(Applausi)*.

molte accertate drammaticamente, altre - ahimè - nemmeno classificate, perché accadono nella notte o nelle acque limitrofe alla Libia. Ci sono tanti martiri ignoti di questa tragedia dell'immigrazione. Se diminuiscono queste tratte (questa tratta e queste tratte di mare), diminuiscono anche le morti. Abbiamo anche intrapreso una politica di realismo. Vedremo se l'esperimento dell'Albania - e dirò da qui a poco qualcosa sulla magistratura ma smettetela di dire bugie. Non è vero che si spende un miliardo. Ha detto il Ministro dell'interno in quest'Aula che, se funzionerà il tutto, si tratta di 160 milioni di euro l'anno. Voi avete speso decine di miliardi con i Governi Gentiloni e Letta per causare un disastro. *(Applausi)*. Decine di miliardi! Sperperatori! Voi avete portato in Parlamento Soumahoro. La vostra politica è stata quella dei parenti di Soumahoro, oggi sotto processo. *(Applausi)*. Noi disprezziamo gli italiani che sfruttano il lavoro nero degli immigrati, ma rileviamo anche che ci sono gli immigrati che sfruttano il lavoro nero dei connazionali, e lo dico sottovoce. Ho letto con orrore la storia di quel lavoratore

di fango per entrare in Parlamento e ne usciranno con la faccia rossa dalla vergogna. *(Applausi)*. Questa è la realtà che noi abbiamo constatato. Questa è la vostra politica.

Quando il Governo ha detto di fare una politica dei respingimenti, anche quella del centro in Albania, la magistratura è insorta come un sol uomo uomo e i giudici hanno detto di no ai rimpatri, ad esempio in Egitto e in Bangladesh. L'Egitto non è un Paese sicuro. Poi c'è stato quello che ha copiato la sua conferenza, che aveva detto in una conferenza che anche la Germania nazista sarebbe stata considerata sicura per quelli che non erano perseguitati ai tempi del nazismo. Poi quella frase che aveva pronunciato in una conferenza un anno fa l'ha rimessa in una sentenza. Io penso che ci siano alcuni magistrati in questo Paese che prima fanno i comizi e poi li trasformano in sentenze, e questo uso politico della giustizia è una vergogna intollerabile. Questo vogliamo dire anche in Parlamento. In Egitto in questo momento, a quest'ora del giorno (sono le ore 11,35 di un giorno di dicembre), ci saranno molti turisti italiani e nelle stagioni più favorevoli ce ne saranno di più. È un Paese sicuro o insicuro? Non deve essere la magistratura a decidere queste cose. Io potrei fare una rapida rassegna dei no dei giudici ai rimpatri in Egitto e in Bangladesh. L'Egitto è un Paese non sicuro, dicono - cito letteralmente - i magistrati; poi tale Musolino, che è un magistrato, dice, giustificando l'uso politico della giustizia: giustizia: «Un magistrato non è un asettico applicatore delle norme. È sottoposto alla legge ma non al potere politico, e non gli è precluso il diritto di manifestare il suo pensiero». E chi lo nega? Ma se il pensiero si fa sentenza, secondo una lettura ideologica e spesso falsa delle norme, siamo all'uso politico della giustizia.

magistratura. Magistratura democratica, nel suo evento celebrativo del sessantennale a Roma, aveva tra i relatori Landini, il quale poi dice che bisogna fare la rivolta; poi non la fa Landini materialmente, ma la fanno Askatasuna e altri centri sociali che feriscono poliziotti e carabinieri, e poi anche a Torino non vengono perseguiti quelli che io vedo al telegiornale, con la faccia scoperta. Si vedono nei servizi giornalistici: non servono i servizi segreti o i reparti speciali per riconoscerli. L'obbligatorietà dell'azione penale, signor Presidente, non viene applicata a quei violenti assalitori della Polizia e spesso sono i giudici che fanno i congressi con Landini che vuole la rivolta sociale. Allora noi non ci fidiamo di Musolino, di Gattuso, di Santalucia, che ogni giorno ci fa sapere qual è il suo pensiero ostile al Governo, o della giudice Albano. Cito quelli che hanno fatto le sentenze più bizzarre in materia di immigrazione. La giudice Albano, una carriera in Magistratura democratica, dice che le intimidazioni contro di lei sono fomentate dal Governo, così come le critiche per le sue frasi politiche e politiciste. Le voglio leggere in Aula, Presidente: l'articolo 12-*bis* dice

Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia». Così resta, oltre che nella legge, anche agli atti degli interventi parlamentari. Poi ci sono Paesi come la Germania o la Svezia che hanno rimandato dei clandestini, e sapete dove? In Iran e in Afghanistan. Io avrei dei dubbi a mandare dei clandestini in un Paese, in Iran, dove ammazzano gli omosessuali, ma nessuno protesta. Quale associazione LGBT va in piazza contro gli *ayatollah* che ammazzano gli omosessuali? che ammazzano gli omosessuali? Nessuna; dopodiché, in altri casi si esprimono. Ma vogliamo parlare dell'Afghanistan? Per la viltà determinata dalle decisioni di Obama del ritiro degli occidentali - perché fu Obama a teorizzarlo e tutto il mondo l'ha seguito - abbiamo abbandonato l'Afghanistan in mano ai talebani. Tuttavia, non vedo, Presidente, cori di sinistra o di femministe in difesa delle donne dell'Afghanistan, a cui si nega il diritto di parlare. Si dice: parlate adesso. Fate una bella manifestazione non violenta insieme a noi per le donne afgane e allora rispetteremo le femministe a fasi alterne, che fanno le femministe in Italia *(Applausi)* e tacciono sulle violazioni che si fanno in alcune parti del mondo. *(Commenti).* Urlate, urlate pure.

perseguitati e si ampliano le quote di ingresso, che questo Governo ha disciplinato, portandole a oltre 400.000 persone l'anno, ossia quasi la popolazione di una piccola Regione italiana

che riguardano anche l'estensione ad anni successivi del cosiddetto decreto-legge Cutro. Si parla di congiungimenti familiari per persone che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, e quindi si disciplinano anche le attività degli ingressi. Insomma, si tratta di un provvedimento ampio, con tanti articoli, che riguarda anche la sicurezza, così come riguarda l'accoglienza, gli ingressi, il lavoro. Questo Governo e questa maggioranza di centrodestra vogliono coniugare la legalità con la giustizia sociale. Questo è un Paese dove c'è il 10 per cento, anche l'11 per cento forse, di popolazione straniera, e non facciamo i razzisti dicendo che, purtroppo, nel numero dei reati… Prima il senatore De Cristofaro ha citato - e ne sono contento - la diminuzione degli omicidi nel nostro Paese. Andiamo però a vedere la statistica dei reati; mentre gli stranieri in Italia sono il 10 per cento, andate a vedere, reato per reato, chi sono chi sono quelli che commettono reati in base alla nazionalità. Non lo voglio dire altrimenti qualcuno si arrabbia, ma andate a vedere nelle carceri la popolazione detenuta e verificate quali sono le nazionalità Noi però accogliamo lo stesso 400.000 persone nella speranza e nella presunzione che daranno risultati il Piano Mattei, gli accordi internazionali e la politica che abbiamo indotto anche l'Unione europea a fare. L'Italia è il confine dell'Europa e anche la von der Leyen, insieme a Giorgia Meloni, è andata a Lampedusa e in Tunisia. C'è chi va in Arabia Saudita a fare soldi e chi resta in Italia per rendere più sicura la nostra Nazione. Per questo votiamo sì alla fiducia e al decreto-legge

Però a Sharm el-Sheikh si sta bene; ci sono tanti posti nel mondo, assolati, con gli ombrelloni, le sedie a sdraio. In realtà non è così. In realtà, dietro tutto questo c'è un fenomeno molto complesso e molto complicato, talmente complicato che non può non può scontrarsi con la piccolezza dell'intervento che abbiamo sentito oggi dal rappresentante del Governo. Non può. Signora Sottosegretaria, tutti gli studiosi del mondo sostengono che le tre principali sfide del millennio siano l'emergenza climatica, la penuria delle materie prime (tra cui l'acqua, che diventerà forse il bene più prezioso), e poi il governo dei flussi migratori. Finalmente la terza sfida epocale, che ci impegnerà in questa nuova era, arriva in Parlamento e voi vi presentate con un decreto-legge. Voi interessate il Parlamento su quel tema, sul quale magari ciascuno di noi può anche pensarla diversamente, citando ad esempio il villaggio turistico di Sharm el-Sheikh, e vi presentate con quindici articoli. Portate in Aula il povero Presidente di Commissione, che dice che non hanno avuto il tempo per esaminare il decreto, e gli dispiace. Ma se non è calpestare la prerogativa del Parlamento questa, quale può essere? Ha ragione il senatore Borghi. Ormai l'abbiamo capito: voi avete un'allergia al confronto, alla discussione, a tutto ciò che è dissenso e tendete in qualche modo a considerarlo una una perdita di tempo. Ma non è così, Sottosegretario. Non è così che si tratta un tema così complicato.

di un tema così delicato, di venire in Aula a dire che non avete avuto il tempo di leggere questo decreto. Altro che Soumahoro! Voi siete moralmente peggio di Soumahoro! E allora io mi domando perché, cosa è successo per vedervi stamattina, Governo e maggioranza, così a testa bassa. Non è che per caso vi siete arresi? Dite la verità: non è che per caso vi siete arresi su quello che era un vostro punto di forza? Sui migranti avete vinto le elezioni. Sui migranti avete promesso l'inimmaginabile. Voi siete quelli che andavate a leggere i cognomi stranieri sui campanelli dei palazzi delle periferie. Non vi arrendete. Non vi arrendete. *(Applausi)*. Avete vinto le elezioni su questo tema, è vero, ma il mese scorso vi sono entrati 8.000 irregolari; solo il mese scorso. Quest'anno ve ne sono entrati irregolarmente 64.000 e l'anno scorso ne sono entrati 120.000. Voi avete battuto e sconfitto il buonismo della sinistra. Siete andati oltre il buonismo della sinistra. Avete battuto il record della sinistra buona e inclusiva. Avete fatto meglio della sinistra.

a noi non importa, noi possiamo anche fermare un Frecciarossa e decidere di scendere per proseguire in macchina, perché tanto a noi gli elettori ci votano lo stesso; noi possiamo fare del Ministero della cultura un luogo di conversazione, di amore, di improvvisazione, perché tanto a noi gli elettori ci votando lo stesso. *(Applausi)*; noi possiamo andare a Rete 4, in trasmissione, e dire che abbiamo alzato le pensioni minime, perché tanto a noi gli elettori ci votano lo stesso. Però attenzione, amici della maggioranza, perché la gente, tra aumento delle tasse, aumento degli irregolari nelle nostre stazioni, nelle nostre metropolitane e nelle nostre periferie; tra aumento delle rapine, dei furti e delle violenze sessuali, così come sono state registrate dal vostro Ministero dell'interno, sta cominciando a farsi delle domande. Attenzione! E la prima domanda che concerne questo decreto è l'Albania, è l'Albania, perché la gente sta cominciando a domandarsi cosa ci fanno quei 300 poliziotti che voi avete portato via dalle nostre periferie e dalle nostre strade per mandarli a custodire una scatola vuota. La gente sta cominciando a farsi questa domanda. Voglio rispondere - per il suo tramite, Presidente - al senatore Gasparri. Che cosa scopriamo in questo testo di 15 articoli scarni e fumosi che non dicono nulla di sostanziale? Scopriamo, all'articolo 12, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, che dobbiamo rifare l'elenco dei Paesi sicuri nella loro interezza *(Applausi)*, e dobbiamo cancellare la frase «di parti del territorio o», che sarebbe Sharm el-Sheik. el-Sheik. Quando chiederete scusa ai magistrati? Oggi dovete chiedere scusa ai magistrati *(Applausi)*, perché oggi, qui, avete scritto che quegli uomini e quelle donne stavano solamente facendo il loro dovere! loro dovere! Avevate scritto un provvedimento che non rispettava quello che avete scritto finalmente stamattina, e cioè la prevalenza del diritto europeo sulla legislazione nazionale; il fatto che un magistrato non può esimersi dal verificare la compatibilità tra le due legislazioni. *(Applausi).* Chiedete scusa per tutto quello che avete detto a quei magistrati in queste settimane! Li avete offesi e insultati. Li avete chiamati i magistrati rossi e adesso siete costretti ad ammettere che avevano ragione! *(Applausi).* Avevano ragione

Vorrei sentire da voi la parola scusa per quello che avete detto in tutte queste settimane. La gente si fa questa domanda: se per caso le zecche rosse, i magistrati rossi non ci fossero stati per il caso Albania, poniamo che

È un tema serio. È un tema maledettamente serio. Ma è più facile prendersela con i magistrati che assumere una posizione di centralità all'interno dell'Unione europea europea o andare in Europa e chiedere un patto di gestione europea che metta in discussione il principio del Paese di primo approdo. È più facile prendersela con i magistrati con i magistrati cattivi, perché quello è complicato; perché magari devi andare a parlare con gli amici del tuo Governo che sono venuti a Pontida e dire loro di prendere le proprie quote al fine di alleggerire i nostri numeri, noi abbiamo il mare e non possiamo costruire muri e fili spinati nel Mediterraneo, e chiedere loro di darci una mano per rendere questo fenomeno condiviso. No, quello è difficile. Il sovranista è bravo quando tu aiuti lui; ma diventa cattivo quando deve essere lui ad aiutare te! vuol dire essere sovranisti. Le scuse sono finite. Signori della maggioranza, signori del Governo, le scuse sono finite, perché adesso al governo dell'Europa ci siete voi, voi, di quell'Europa cattiva, di quell'Europa tecnica dei burocrati. No, siete diventati voi adesso Europa e potete fare quello che volete, perché state dicendo che siete entrati nella centralità della *governance* europea, avete anche un vicepresidente. allora stare le scatole vuote buttate in Albania, chiudete tutto, riportate i poliziotti e i carabinieri qui in Italia che ne abbiamo bisogno. Lasciate perdere i magistrati e andate in Europa e fate presente che i fenomeni migratori non si possano disciplinare con dieci paginette di decreto-legge, come avete fatto qui, ma ci vuole una discussione allargata e partecipata di tutta l'Unione europea. Questo dovete fare, se siete capaci; altrimenti andate in vacanza a Sharm el-Sheikh e che Dio vi benedica.

partendo dal quello del collega che mi ha preceduto, affermando che anche noi rispettiamo pienamente l'operato dei magistrati che applicano la legge,

Dico anche che il nostro Gruppo voterà questa fiducia convintamente, perché è un atto di fiducia nei confronti di un Governo che sta gestendo bene il tema dell'immigrazione.

che le politiche del Governo e le leggi approvate in Parlamento da questa maggioranza hanno un'efficacia reale e concreta.

Anche da questo punto di vista, se fosse giusta la vostra teoria, dovremmo avere dei numeri in decrescita, come se noi fossimo ideologicamente contrari agli immigrati, all'immigrazione regolare, con cui si cercano lavoro e opportunità e si dà sviluppo al nostro Paese. i numeri vi danno torto, perché nel provvedimento in discussione si parla di un aumento significativo degli ingressi regolari dei lavoratori stagionali di oltre

questa parte rilevante della nostra economia. Ciò, altresì, a dimostrare che non c'è alcun pregiudizio nei confronti degli immigrati che vogliono lavorare e dare sviluppo al nostro Paese.

analisi dettate dalle evidenti differenze che esistono tra noi e voi. Innanzitutto, una delle critiche emerse è legata al fatto che in due anni abbiamo portato avanti troppi provvedimenti sul tema dell'immigrazione: otto decreti-legge. sé, questo non è un problema, non significa che non abbiamo le idee chiare sull'immigrazione. Significa esclusivamente che, a fronte di leggi approvate, abbiamo anche la capacità di intervenire per migliorarle, per adattarle alle circostanze che cambiano, con la volontà che siano le più efficaci possibili e abbiano una durata che

una legge quadro sul tema dell'immigrazione che è stata citata più volte. Esiste la legge Bossi-Fini, approvata dal centrodestra nel 2002,

Prodi ai Governi Letta, Gentiloni e Renzi, fino al Governo Conte, appoggiato dal MoVimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Italia Viva. Avete avuto più occasioni di abrogare questa legge, che per voi è foriera di chissà quali danni al nostro Paese. Non l'avete fatto e quindi si dimostra tutta la vostra ipocrisia, o forse anche la realistica convinzione che, tutto sommato, quella legge non è poi così male come la descrivete quando siete all'opposizione. *(Applausi)*. Le differenze tra noi e noi riteniamo che l'immigrazione vada regolamentata, che servano regole, che non possa passare il principio che chiunque possa varcare i confini senza controllo e verifica dei requisiti. Questa non è xenofobia, non è razzismo, ma è la volontà di dare ordine a una materia molto complessa. Questi fenomeni sicuramente non possono essere arrestati completamente, ma proprio perché sono così invasivi e importanti vanno gestiti. Ricordo al senatore Renzi che forse l'apice dell'improvvisazione

perché non ragioniamo come voi, non come un Governo di sinistra. Poi c'è il tema della sicurezza. Voi continuate a ritenere che non esista una correlazione tra immigrazione incontrollata e sicurezza. Noi abbiamo una visione totalmente diversa. Come abbiamo sentito anche da esponenti intervenuti in queste dichiarazioni di voto, non esiste un problema sicurezza ed esistono situazioni di insicurezza ben superiori in Gran Bretagna e Francia. a parte che a noi non interessano questi confronti, ma interessa il dato reale dell'Italia che sta peggiorando di anno in anno, osservo che i livelli di insicurezza raggiunti in quei Paesi derivano in gran parte proprio dall'immigrazione.

è il *trend*. Che esista una correlazione lo dicono sempre i numeri, che non possono essere controvertiti dalle parole. Sappiamo quello che è avvenuto a Milano, con la rivolta innescata da gruppi incontrollati di immigrati, e sappiamo quanto ha dichiarato il ministro Piantedosi, che ha riferito che in quell'area i reati legati alla presenza degli immigrati è pari al 65 per cento del totale dei reati commessi. Mi sembra che il dato sia significativo e preoccupante. Questo dato riguarda una grande città, città, una grande metropoli italiana, ma il fenomeno, purtroppo, rischia di dilagare in ogni nostra città. Vediamo di giorno in giorno, di anno in anno, quanto le nostre città stiano diventando sempre più insicure. A questa affermazione e a questa nostra visione delle cose voi rispondete con il concetto della scorretta percezione della sicurezza, come se quello che sentono, vedono e vivono i cittadini italiani sia falso e frutto di propaganda politica. Potete dirle queste cose, ma ogni cittadino italiano sa che la sicurezza nella propria città sta peggiorando di anno in anno e che purtroppo il fenomeno immigratorio incontrollato, quando non è regolamentato, è un fattore che incrementa questo stato di insicurezza. sono poi delle teorie che io non condivido. La vostra teoria è che l'immigrazione è la soluzione a tutti i problemi. Ci sono meno figli?

è un problema che va affrontato anche e soprattutto con aiuti alle famiglie italiane per fare più figli, che siano aiuti sia economici, sia fiscali. Apprezzo molto che questo Governo,

di quella che per noi è la linea da seguire per combattere il fenomeno della denatalità. Non è certamente con la sostituzione dei figli degli italiani con persone che provengono da altri Paesi che si dà risposta a questo fenomeno.

l'interprete di governo che ha combattuto il fenomeno dell'immigrazione clandestina con più efficacia, coraggio e determinazione e proprio per questi motivi oggi è sotto processo per sequestro di persona. *(Applausi)*.

intollerabile che un Ministro che compie il proprio dovere sia oggi sotto processo per reati che non esistono, come il sequestro di persona, per aver trattenuto in mare

situazione tutta italiana, in cui la sinistra, non riuscendo a sconfiggere gli avversari nelle urne, a volte - anzi, spesso - ha la tentazione di ritenere legittimo farlo nelle aule dei tribunali. *(Applausi)*. Noi non apprezziamo questo modo di di affrontare il confronto politico e con coraggio e determinazione portiamo avanti le battaglie contro l'immigrazione clandestina e a favore dei flussi regolari, convinti che questo Governo stia percorrendo la strada giusta. Per questo motivo, anche quest'oggi daremo il nostro voto di fiducia. *(Applausi)*.

anche attraverso un'interlocuzione serrata col Governo, di valutare con cura gli effetti di ciascuna delle molteplici ed eterogenee disposizioni e di risolvere le molte contraddizioni e i profili di inefficacia e di dubbia legittimità che emergono fin da una primissima lettura.

Eppure, onorevoli colleghi, di discutere e di approfondire ce ne sarebbe stato un gran bisogno, perché non riusciamo davvero a comprendere quali siano i benefici, per il nostro Paese, il nostro sistema produttivo e la sicurezza dei cittadini, che derivano dal perseverare, come fate anche con questo decreto, nell'escludere, da un lato, ogni regolarizzazione di coloro che sono già presenti sul territorio e, dall'altro, nello stabilire quote di ingresso regolare del tutto insufficienti a soddisfare la domanda di forza lavoro che proviene da diversi settori produttivi, dal settore manifatturiero a quello agroalimentare e a quello turistico. Il principale effetto di questo indirizzo sarà quello di aumentare il numero delle presenze irregolari, alimentare lo sfruttamento e il lavoro nero e, al tempo stesso, accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità. Altro che tutela della sicurezza, altro che sostegno alle imprese che rispettano le leggi, altro che contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Non molto dissimile temo che sia l'effetto della disposizione che esclude i patronati dal novero dei soggetti che sono abilitati a inviare le richieste di ingresso e di nulla osta al lavoro un servizio e un'assistenza gratuita che si sono dimostrati preziosi ed aumenterà così il rischio, per molti richiedenti, di non riuscire a rispettare i tempi già molto compressi per la presentazione delle domande e dunque aumenterà il rischio di scivolare nell'irregolarità. E quali effetti positivi dovrebbero discendere, colleghi, dall'ostacolare i ricongiungimenti familiari, raddoppiando gli anni di permanenza continuativa e incrementando i requisiti per avanzare la relativa richiesta, a partire dalla disponibilità di un alloggio conforme a determinate caratteristiche igienico-sanitarie e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali, che chi richiede il ricongiungimento dovrà farsi rilasciare? Chi di voi pare rendersi conto della necessità di una nuova e più moderna disciplina della cittadinanza, imperniata sul criterio dello *ius soli* o dello *ius e comunque propone di riconoscere fin da subito la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri e chi di voi predica la centralità della famiglia e dei relativi legami come può votare a favore di una disposizione che muove nella direzione esattamente opposta? *(Applausi)*. Come può approvare una disposizione che avrà come unico effetto quello di aumentare la sofferenza e la solitudine e di ostacolare la volontà di integrazione e di appartenenza alla nostra comunità? dopo la tragedia che si è consumata presso le coste di Cutro e dopo le morti in mare che si sono susseguite, ci saremmo attesi delle misure per garantire un più coordinato ed efficace intervento di soccorso e per provare a rimuovere le cause di viaggi pericolosi e in condizioni inumane e degradanti; invece, sul punto troviamo solo norme che mirano ad ostacolare ulteriormente l'opera di soccorso delle ONG.

se l'immigrazione diminuisse, il rapporto debito-PIL salirebbe e anche in maniera significativa. E allora perché non abbandonare questa prospettiva ottusa e meramente repressiva? Perché non avviare un confronto pubblico vero, aperto, coinvolgendo gli amministratori locali e facendo tesoro delle loro competenze e delle loro esperienze *(Applausi)*, insieme a quelle dei molti che operano nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione, spiegando innanzitutto ai cittadini che non è vero che «ogni L'espressione è di Primo Levi, che metteva in guardia sulle conseguenze del diffondersi di una simile convinzione. Ogni straniero è innanzitutto una persona titolare di diritti e di doveri, come ogni essere umano, ed è una potenziale risorsa per l'intera collettività. Certo, la convivenza tra persone che hanno culture, tradizioni ed esperienze diverse è più difficile e più impegnativa, richiede investimenti culturali ed economici, ma alla fine è anche la strada più efficace per garantire sicurezza e promuovere crescita e sviluppo. siamo pronti a fare la nostra parte, con convinzione e responsabilità. Ecco, di questo avremmo voluto discutere nel corso dei lavori parlamentari: di come affrontare un fenomeno strutturale ed epocale, qual è l'immigrazione, in maniera efficace e rispettosa dei princìpi costituzionali e del diritto internazionale, senza cedimenti alla demagogia. Ma non è stato possibile: non lo ha consentito il Governo e non lo consentite voi, senatori della maggioranza, che accettate di trasformarvi da legislatori in meri esecutori di scelte politiche e normative che vengono definite altrove. Governo, infatti, senza che peraltro sussistesse alcuna situazione straordinaria di necessità e urgenza, ha adottato l'ennesimo decreto-legge per disciplinare l'ingresso dei lavoratori stranieri, il cosiddetto decreto flussi. Poi ha adottato un secondo decreto-legge, anche in questo caso senza che vi fosse alcuna situazione straordinaria di necessità e urgenza, per disciplinare le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e, in particolare, per definire i cosiddetti Paesi sicuri. Poi ha fatto confluire il secondo decreto-legge in un emendamento alla legge di conversione del primo, riducendo così ulteriormente i tempi a disposizione del Parlamento per la discussione; tempi che al Senato sono venuti del tutto meno, tant'è che in Commissione non è stato discusso neanche un emendamento. Ora, che un simile modo di legiferare violi le più fondamentali prerogative del Parlamento è indubbio. La sottoposizione delle Camere al Governo è totale. Ma in questo caso si è consumato anche il tentativo di sottoporre al Governo la magistratura, di aver fatto prevalere sulla volontà del Governo il diritto europeo e alcuni princìpi costituzionali che disciplinano il nostro sistema delle fonti. Che cosa è accaduto? è accaduto? Diversi tribunali, facendo prevalere il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di giustizia, hanno disapplicato parte del decreto interministeriale con cui il Governo aveva definito l'elenco dei Paesi di origine sicuri. In particolare, non hanno convalidato il trattenimento di alcuni migranti che erano stati sottoposti alla cosiddetta procedura semplificata, sul presupposto che provenissero da Paesi sicuri. A questo punto il Governo, anziché conformare la propria azione alle pronunce dei tribunali e a quanto disposto dalla Corte di giustizia, ha pensato di potersi sottrarre ai limiti del diritto europeo elevando il rango della propria disciplina e ha così trasferito il contenuto del decreto interministeriale in un decreto-legge. Naturalmente ciò non ha consentito al Governo di superare alcun limite posto dal diritto europeo e dalla nostra Costituzione ed applicato dai tribunali, perché anche la legge e il decreto-legge sono gerarchicamente subordinati al diritto europeo e alla Costituzione. Quindi, com'era prevedibile, i tribunali hanno disapplicato anche parte del suddetto decreto-legge e hanno rimesso la questione alla Corte di giustizia. allora il Governo? Con un ulteriore emendamento, battezzato con una certa efficacia «emendamento Musk», ha tolto la competenza ai tribunali, in particolare alle sezioni specializzate che erano state appositamente create per trattare questa delicata e complessa materia, e l'ha trasferita alle corti d'appello in composizione monocratica, arrecando in tal modo un danno significativo anche all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari di secondo grado (danno che i presidenti hanno infatti subito denunciato). emerge in questa vicenda un tratto politico e culturale che è tipico dell'azione di questo Governo e delle forze politiche che lo sostengono, che si potrebbe sintetizzare nell'avversione al pluralismo - e quindi al Parlamento quale luogo di rappresentanza e composizione del pluralismo politico e sociale - e a ogni limite al potere della maggioranza in nome di una concezione illiberale ed autoritaria della democrazia, ovvero in nome di una omogeneità e di un ordine ideali, che la maggioranza, in quanto tale, pensa di avere il diritto di imporre, superando, se necessario, ogni limite posto dalla Costituzione o dal diritto europeo. Il tutto, accompagnato da una spregiudicatezza politica che, per conquistare un po' di consenso immediato, non si fa scrupoli di far leva sulle paure e sulle pulsioni più irrazionali e distruttive. Onorevoli colleghi, credo che voi stiate sottovalutando l'umanità, la saggezza e l'intelligenza dei nostri concittadini e penso che di fronte agli evidenti insuccessi delle vostre politiche, del centro costruito in Albania, non ci sia più nulla da aggiungere, se continuerete solo a paventare il rischio dell'invasione…

*(PD-IDP)*. Di fronte agli evidenti insuccessi delle vostre politiche, se continuerete solo a paventare il rischio dell'invasione, a inasprire la dimensione meramente repressiva e a denunciare l'illegittimità dell'azione della magistratura, che si permette di far valere alcuni fondamentali principi giuridici e di civiltà, alla fine gli elettori vi puniranno, perché vedranno solo aumentare la sofferenza, la paura e l'esclusione sociale e non certo la sicurezza e la qualità della loro vita. Per queste ragioni voteremo contro la conversione in legge dei due decreti, ma rimarremo disponibili a un vero e aperto confronto nell'interesse del Paese e di una convivenza rispettosa dei principi di uguaglianza e di libertà sanciti dalla Costituzione e dal diritto europeo e internazionale.

il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo disegno di legge di conversione, perché siamo determinati a sconfiggere l'immigrazione illegale. *(Applausi)*. È un impegno che abbiamo preso con gli italiani, che ci hanno dato fiducia anche per questo. Siamo determinati a sconfiggere l'immigrazione illegale, perché crediamo che chi deve venire in Italia lo debbano decidere le autorità, lo Stato, il Governo e non gli scafisti e i mercanti di esseri umani. Anche per questo abbiamo aumentato a 452.000 ingressi regolari i flussi in tre anni, numeri che oggi voi criticate, ma ai quali non vi siete nemmeno lontanamente avvicinati negli anni in cui potevate farlo, visto che siete stati al Governo quasi ininterrottamente dal 2011 al 2022, con una piccola parentesi.

che a favore dell'immigrazione selvaggia, incontrollata e senza regole militano fortissimi interessi. Sappiamo bene quali sono questi interessi: nel *business* più remunerativo della nostra epoca, più del traffico di droga e di quello di armi. Quindi, certo, abbiamo come nemici prima di tutti gli scafisti,

le cooperative, i patronati, i sindacati, tutte che le associazioni che lucrano su quella cifra di 1,8 milioni di euro che ogni anno l'Italia destina all'accoglienza. Se venisse meno l'immigrazione irregolare, tanti di costoro dovrebbero cercarsi un altro lavoro. E che dire di certe ONG che hanno trasformato il soccorso in mare in un lavoro ben remunerato. Ogni riferimento allo stipendio che Casarini si è autoliquidato è puramente voluto, ovviamente. *(Applausi)*. abbiamo tutti questi grandi e grossi interessi contro e sappiamo anche che (si potrebbe parlare di convergenze parallele con tutti questi attori che ho appena nominato) abbiamo anche l'attore più forte e più importante di tutti questi, che insieme a loro lavora nella stessa direzione, cioè la sinistra. La sinistra sa bene che sul tema dell'immigrazione il centrodestra ha preso un impegno preciso con gli italiani e fa di tutto per sabotare. Abbiamo sentito anche molti interventi. Fino Fino a poco tempo fa parlavate di redistribuzione. Adesso che anche Scholz, Macron, e Starmer vi danno torto, avete ripiegato sulla regolarizzazione: voi volete regolarizzare tutti i clandestini che abbiamo in casa. Quando eravate al Governo, li volevate espellere: avete fatto la legge sui CPR, salvo poi sabotarla nel momento in cui non siete stati più al Governo e denunciarla come un abominio.

la politica contro le porte aperte e l'immigrazione indiscriminata, che voi con le vostre leggi (vedi il cosiddetto decreto Lamorgese) avete favorito. con il decreto Lamorgese avete scritto a caratteri cubitali in tutto il Terzo mondo: venite in Italia perché chiunque riuscirà a mettere piede in Italia ci potrà rimanere. vi meravigliate del fatto che nel 2022 sono arrivati 150.000 migranti in un anno solo? Ci mancherebbe, avete lavorato dieci anni per ottenere questo risultato. Complimenti, ci siete riusciti.

Si dà il caso, ad esempio - a voi dispiace, lo so -, che soltanto quest'anno, grazie agli accordi che ha concluso il Presidente del Consiglio insieme all'Unione europea… si può lamentare a correnti alternate. Stavo dicendo - sono dati ufficiali - che soltanto quest'anno, grazie agli accordi che ha concluso il presidente del Consiglio italiano, onorevole Giorgia Meloni, insieme al Presidente della Commissione europea, con la Tunisia e con altri Paesi rivieraschi,

fermati; non sono arrivati perché non sono partiti o, se sono partiti, sono stati bloccati e riportati indietro. Nessuno mi toglierà dalla testa che 100.000 partenze in meno vuol dire anche migliaia di morti annegati in meno. Questo grazie al Governo Meloni. Fosse stato per voi, quest'anno non sarebbero arrivati 63.000 migranti con gli sbarchi, ma ne sarebbero giunti 163.000, ed è esattamente quello che avreste voluto. Quindi capisco perché vi state battendo anche contro la conversione di questi decreti-legge. Non basta. Dicevo che quest'anno sono arrivati 63.000 migranti, 90.000 in meno dell'anno scorso

che non è arrivata in Italia e meno possibilità di lucrare su tutta la filiera dell'accoglienza. Lo so che vi brucia, ma questa è la realtà. Basta? Non basta, perché certamente, con le misure che oggi variamo, otterremo ulteriori risultati. Misure che - ve lo segnalo sommessamente vanno anche contro il caporalato (non ho sentito una parola da parte vostra), vanno contro chi sfrutta gli immigrati irregolari (non ho sentito una parola da parte vostra), vanno a difesa dei testimoni che decidono di denunciare (non ho sentito una parola

Come tutti sappiamo, la sentenza della Corte europea del 4 ottobre, a cui continuate a fare riferimento, vi ha spiegato anche il giudice emerito della Corte penale internazionale Cuno Jakob Tarfusser,

definire sicuro un Paese soltanto limitatamente a una porzione del suo territorio. Il caso giudicato, come sappiamo, la Moldavia in relazione alla Transnistria, che è sotto il controllo dell'occupante russo. Ma nulla ha detto in relazione alle condizioni soggettive di determinate categorie: perseguitati politici, *gay* e via di questo passo. In relazione a questo, autorevoli giuristi sostengono che non è possibile per il giudice italiano entrare nel merito. Lo ha detto anche una sentenza della Corte di cassazione del 27 settembre (andatevela a leggere).

Quindi non è possibile che un giudice ignori la lista dei Paesi sicuri. Se un Paese è definito sicuro, il giudice ne deve prendere atto, salvo, con inversione dell'onere della prova, che sia il soggetto interessato a dare prova, in concreto, di appartenere a una determinata categoria soggettiva per la quale avrebbe comunque diritto alla protezione internazionale. La dice che c'è un'inversione dell'onere della prova. Ebbene, nelle sentenze dei giudici dei tribunali italiani che hanno disapplicato la normativa italiana sulla scorta di una sentenza della Corte europea che diceva tutt'altro, come vi ho appena dimostrato, non c'è una sola riga in cui si dimostra che quel determinato soggetto appartiene a una categoria che soggettivamente meriterebbe la protezione. Il giudice italiano si è cioè arrogato il diritto di stabilire, non si sa sulla base di quali informazioni e criteri, se un Paese è sicuro oppure no. Non si può fare, tant'è vero che, anche dopo l'emanazione di questo decreto-legge, i giudici più avveduti si sono guardati bene dal disapplicare la normativa. Si sono limitati - e questo è legittimo - a rivolgersi alla Corte europea per chiedere se è legittimo o meno estendere le condizioni oggettive anche a determinate situazioni soggettive. C'è chi dice che si può, c'è chi dice che non si può, io non ho la verità in tasca. Prendo tuttavia atto, chiunque abbia ragione, che stiamo discutendo soltanto di pochi mesi perché tutti sappiamo che nella primavera del 2026 entrerà in vigore il nuovo patto per la regolamentazione di questa materia, che prevede una disciplina esattamente corrispondente a ciò che sta

tranne il PD, che è rimasto indietro anche rispetto ai suoi colleghi europei. Per tutte queste ragioni, il Gruppo Fratelli d'Italia esprimerà un voto convintamente favorevole.

dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: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

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Berrino.

Dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1310, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145,

apre una nuova finestra") ***Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione*** ***se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo all'utilizzo di videoregistrazioni effettuate da un privato nell'ambito di un procedimento penale

in quanto l'autorità giudiziaria non ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003. La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Domando al relatore, senatore Maffoni se intende integrare la relazione.

per intercettare un parlamentare o registrare un parlamentare occorre ovviamente rispettare la Costituzione e quindi avere l'autorizzazione della Camera di

Saremmo al paradosso per cui il privato può raggiungere un risultato che nemmeno le Forze dell'ordine possono ottenere senza passare attraverso l'autorizzazione delle Camere.

interverrò molto brevemente perché credo che il relatore Balboni abbia spiegato il punto fondamentale di questo caso. Come sappiamo, l'articolo 68 della Costituzione prevede che per intercettare i membri del Parlamento

senza che il senatore Giovanardi lo sapesse, e queste registrazioni sono state usate in giudizio. È evidente che se la Costituzione richiede che le intercettazioni siano autorizzate, comunque esse siano fatte e da chiunque siano fatte, è chiaro che il tribunale di Modena, non richiedendo l'autorizzazione al Senato,

stiamo assistendo alla creazione di fatto di una immunità non più soltanto funzionale, quindi indissolubilmente legata allo svolgimento delle funzioni del parlamentare, bensì di fatto sostanzialmente personale, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Unitamente a ciò, assistiamo a costruzioni logiche fuorvianti e prive di ragionevolezza, volte ad assoggettare gli strumenti che offre l'ordinamento giuridico al precipuo fine di garantire comunque l'effetto impeditivo conseguente alla delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera di appartenenza del parlamentare. La Corte costituzionale, Presidente, si è già pronunciata sul caso Giovanardi: i fatti esulerebbero completamente dalla prospettiva di critica e denuncia politica e non presenterebbero alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, trattandosi di condotte rivolte direttamente agli organi competenti e ai loro componenti, al fine specifico di ottenere la modifica puntuale di singoli provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese dallo stesso indicate. una pronuncia così incontrovertibile, cosa fa la Giunta e di cosa siamo testimoni, sempre in Giunta? Ripropone un conflitto di attribuzione, lo stesso stratagemma utilizzato nella passata legislatura e poi abbandonato abbandonato per utilizzare la strada della pronuncia di insindacabilità, stroncata dalla Consulta. Anche in questo caso la soluzione scelta non appare percorribile, in quanto il costrutto logico-giuridico che attiene all'equiparazione tra videoregistrazioni e intercettazioni non ci convince. Non vi è traccia nell'ordinamento di quanto affermato nella relazione conclusiva. Nessuna disposizione normativa prevede l'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per l'utilizzo, nei confronti di un parlamentare, di videoregistrazioni effettuate da privati. Se la normativa non lo prevede, la giurisprudenza della Cassazione addirittura lo esclude, ricomprendendo infatti le videoregistrazioni nella categoria delle prove documentali di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale, in cui sono ricomprese le rappresentazioni di fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (quindi anche le videoregistrazioni). Per queste ragioni, le richieste e le deduzioni del relatore

il procedimento Giovanardi è un caso di cui ci siamo occupati frequentemente, anche nella passata legislatura, laddove questa Assemblea aveva Assemblea aveva votato originariamente contro una relazione sulla sindacabilità del relatore originario, per poi votare per un'insindacabilità su tutti i profili che erano stati contestati. Successivamente la Corte ha in realtà deciso in senso conforme alla relazione dell'epoca, che era stata del senatore Durnwalder. Ma noi oggi discutiamo di un'altra questione, quella di sollevare un conflitto di attribuzione su un profilo che obiettivamente è giuridicamente interessante. Cosa è successo rispetto alla passata legislatura? Nella scorsa legislatura,

non era processualmente venuta in essere una richiesta di utilizzazione di quello di cui oggi stiamo discutendo, ovvero - come è stato citato nella relazione del senatore Balboni - una videoregistrazione tra privati. Adesso invece questa utilizzazione è venuta all'evidenza. Perché dico che è interessante? Perché in questi ultimi anni si sono verificati una serie di fatti. Il primo fatto è che i mezzi a disposizione di chiunque per registrare o videoregistrare sono diventati tantissimi. Era impensabile, quando sono state scritte una serie di norme, che fosse così facilmente utilizzabile un mezzo per registrare o videoregistrare. Il secondo fatto che è intervenuto è che c'è stata un'evoluzione della giurisprudenza, anche costituzionale, che muove dal fatto che il tenore letterale dell'articolo 68 sembrerebbe individuare e perimetrare il concetto di intercettazione di comunicazioni, conversazioni o corrispondenza in un modo molto ampio, nel senso che usa l'espressione «in qualsiasi forma». D'altra parte, il susseguirsi di una serie di pronunce della Corte di cassazione e della stessa Corte costituzionale, quando ha fatto rientrare in questo concetto, per esempio, i tabulati, ribadendo che sono coperti dalla prerogativa per cui è necessario chiedere l'autorizzazione anche per essi e non soltanto per le intercettazioni di

queste prerogative sono a garanzia del non condizionamento del Parlamento e, quindi, in questo senso del singolo parlamentare. A me piace sottolinearlo perché in questo caso, come in altri casi, non discutiamo di un regime diverso e in qualche modo privilegiato: stiamo discutendo delle garanzie e delle prerogative del Parlamento. Parlamento. In concreto che cosa potrebbe succedere oggi in assenza di un intervento legislativo chiarificatore? Laddove interviene l'autorità giudiziaria, ci sono una serie di garanzie - deve essere chiesta l'autorizzazione prima o comunque dopo per l'utilizzo - viceversa, se vi è una registrazione o videoregistrazione da parte del privato, privato, rientrerebbe nella disciplina che per prassi viene adottata e viene assimilato in tutto e per tutto a un documento e, in quanto tale, verrebbe acquisito senza necessità di autorizzazione.

che il dubbio è assolutamente legittimo. C'è un vuoto legislativo che non tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza, del tenore dell'articolo 68 e di quello che in concreto oggi si può verificare e in passato non era neanche lontanamente immaginabile.

sostanzialmente è il mezzo stabilito quando c'è stata effettivamente un'esondazione. In tal caso più che di esondazione, possiamo dire che

collettiva e laica, anche con un'iniziativa del legislatore su tutti questi punti nel mondo che cambia.

il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003. *(Segue la votazione).*

Allegato B)*. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla perquisizione domiciliare, all'utilizzo di intercettazioni ambientali, nonché di filmati di videosorveglianza, effettuati dall'autorità giudiziaria nei locali della segreteria politica dell'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti,

procedente non ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte della Camera competente, in violazione all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Signor Presidente, come nel caso precedente, noi voteremo a favore del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Lo faremo per riaffermare la vigenza dell'articolo 68 della Costituzione, in base al quale i componenti del Parlamento, deputati e senatori, non possono essere intercettati in qualsiasi forma Non possono essere perquisiti il loro domicilio e la loro persona non in senso assoluto,

o alla senatrice, ma che per preservare la libertà del mandato parlamentare, cioè la rappresentanza del corpo elettorale che ci ha mandato qui, la Camera di appartenenza deve verificare se la richiesta di perquisizione o di intercettazione sia motivata, per esempio, da *fumus persecutionis.* Questa non è una bizzarria della Costituzione, che si è ispirata al principio della separazione dei poteri, per cui, per esempio, quest'Assemblea non discute di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, né ne stabilisce il trasferimento di ufficio, perché la magistratura ha un organo di autogoverno. Allo stesso modo la funzione legislativa deve essere preservata da eventuali situazioni che possano configurare un *fumus persecutionis.* Lasciatemi ricordare in quest'Aula i sette anni passati dal nostro ex collega Stefano Esposito, che è stato sottoposto a un'indagine, archiviata con molte scuse e basta, dopo che una reputazione e una carriera politica sono state distrutte. Ricordo, peraltro, che l'archiviazione è stata richiesta dalla procura della Repubblica di Roma, quindi dalla pubblica accusa. Ebbene, questo rafforza la convinzione che l'articolo 68 stia bene dov'è e che vada applicato nella sua integrità. Dico ai colleghi dei Gruppi politici che votano costantemente contro l'articolo 68: dato che avete il potere di iniziativa legislativa, depositate un disegno di legge costituzionale che abroghi l'articolo 68. Però, finché l'articolo 68 è 68 è parte della Costituzione cosiddetta più bella del mondo, io proporrei a quest'Aula di rispettare l'articolo 68. L'articolo 68 dice che, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, un parlamentare non può essere né intercettato né perquisito. Nel caso precedente parlavamo delle intercettazioni surrettizie, clandestine quasi, fatte da un terzo a carico del senatore Giovanardi. Qui parliamo della perquisizione degli uffici della collega Sudano, attualmente deputata, all'epoca dei fatti senatrice. Era di dominio pubblico che quelli fossero gli uffici di un parlamentare e l'autorità giudiziaria, quindi, non ha rispettato l'articolo 68. Ribadisco il concetto. Noi stiamo proponendo di sollevare un conflitto d'attribuzione davanti alla Corte perché, nonostante la vigenza dell'articolo 68, le due autorità giudiziarie, nel caso precedente il tribunale di Modena e in questo caso la procura di Catania, hanno ignorato l'articolo 68 e intercettare. Avrebbero potuto comunque procedere. Sarebbe bastato chiedere alla Giunta presieduta dal collega, presidente Franceschini, l'autorizzazione a farlo, così come la Costituzione. Invece, sono andati avanti senza l'autorizzazione e quindi mi pare ovvio che noi chiediamo alla Corte costituzionale di difendere le prerogative del Parlamento; così come sarebbe legittimo che la magistratura chiedesse di difendere le sue prerogative, se noi improvvisamente in quest'Aula iniziassimo a trasferire magistrati o a stabilire sanzioni disciplinari: cosa che naturalmente ci guardiamo bene dal fare. Quindi, indipendentemente dalle figure politiche di cui stiamo parlando, dalla loro storia, dalle loro opinioni, delle quali poco ci interessa in questo caso, noi dobbiamo limitarci a rispettare la Costituzione - cosa che abbiamo tutti giurato di fare - e applicare, fintanto che è vigente, l'articolo 68, la cui lettera mi pare molto chiara.

in violazione dell'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare,

recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***

Signora Presidente, l'articolo 1 torna sulla disciplina delle valutazioni ambientali, più volte modificata nel corso degli ultimi anni.

Durante l'esame in Commissione sono state apportate varie modifiche. Si è tra l'altro previsto che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale a ciò finalizzato, siano da considerarsi prioritari anche: i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi d'acqua immagazzinabili; le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi agli impianti industriali oggetto di conversione; di conversione; i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 megawatt. Viene differita al 30 giugno 2026 la possibilità di ricorrere alla videoconferenza per i compiti istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle sottocommissioni e dei gruppi istruttori. La possibilità di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale dell'Arma dei carabinieri è estesa anche alla commissione PNRR-PNIEC, e ad entrambe le commissioni è riconosciuta la possibilità di avvalersi inoltre di quattro unità di personale del Corpo della guardia di finanza. Si prevede che, tra i documenti allegati dal proponente all'istanza di VIA, vi debba essere anche un'autodichiarazione relativa agli assetti proprietari della società proponente e dell'eventuale società controllante, e alla consistenza del capitale sociale della società proponente. [**Presidenza del vice che, per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare, termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA alleghi una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto,

Il comma 4 autorizza il Ministero della difesa a definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti delle infrastrutture e dei beni del demanio militare. Qualora il programma o i singoli interventi in esso inseriti siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del codice dell'ambiente, tali procedure sono svolte dalla commissione PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. Le medesime misure di semplificazione trovano applicazione, ai sensi del comma 5, con riferimento agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa. L'articolo 2, comma 1, abroga le disposizioni che disciplinano il Piano per la transizione energetica delle aree idonee (Pitesai)

in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è stato recentemente annullato dal TAR del Lazio. Il comma in esame riconosce, inoltre, il carattere di pubblica utilità delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, già previsto nel 2014 e poi disapplicato dalla stessa normativa che ha introdotto il Pitesai. Il comma 2 vieta il conferimento di nuovi permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fatta eccezione per le concessioni da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi già rilasciati. Le attività di coltivazioni svolte sulla base di concessioni già conferite o che possono ancora essere conferite nei termini predetti proseguono per la durata di vita utile del giacimento. Il comma 3 concerne le proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi al fine di tararle sul tempo effettivamente necessario per la messa in produzione delle riserve accertate, con possibile riperimetrazione di aree non necessarie da poter ridestinare, dunque, ad altri usi. Il comma 4 riduce da 12 a 9 miglia dalla linea di costa e dalle aree protette il perimetro dell'area in cui vige il divieto di svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di Il comma 5 interviene sulla disciplina del *gas release*, prevedendo che nell'alto Adriatico sia consentito, ai soli fini della partecipazione alla procedura in questione, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate, a patto che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. La relazione illustrativa chiarisce che è una sola l'istanza già presentata che rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disposizione in esame. La Commissione ha apportato modifiche al comma 6, che interviene sulla disciplina del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi, prevedendo che il termine ultimo della vendita e le relative modalità siano stabiliti con atto di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire la massima flessibilità a beneficio del sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE per il nuovo anno termico. Viene conseguentemente posticipato al 10 dicembre 2027 il termine per la restituzione del prestito.

l'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di gestione della crisi idrica. La lettera *a)* del comma 1 introduce una nuova definizione di acque affinate, che include, oltre alle acque urbane, le acque reflue domestiche e industriali. La lettera chiarisce i casi in cui le Regioni non violano la normativa in materia di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque all'avverarsi di un deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici idrici e prevede che esse comunichino tempestivamente alle Autorità di bacino le misure adottate al fine di conservare lo stato qualitativo dei corpi idrici. La lettera *c)* contiene una modifica di coordinamento, la lettera *d)* prevede che il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei possano essere autorizzati non solo al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dei corpi idrici, ma anche in caso di crisi idrica, e che essi possono essere effettuati impiegando anche le acque affinate, come definite dalla precedente lettera *a)*. La lettera *e)* amplia la definizione di servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque Il comma 2 autorizza il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane a esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi della risorsa stessa. I commi 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti nel corso dell'esame in Commissione, dettano disposizioni relative alla società Acquedotto Pugliese SpA. In particolare, il comma prevede che almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società siano designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della rilevanza strategica per l'interesse nazionale dell'attività svolta dalla società stessa. Il comma 2-*ter*, al fine di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità della gestione *in house*, autorizza la Regione Puglia a trasferire parte delle azioni della società in favore dei Comuni della medesima Regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per la finalità di cui all'articolo 149-*bis* del testo unico ambientale ovvero in favore di quest'ultima società. L'articolo 4, comma 1, prevede che il gruppo di lavoro incaricato di svolgere le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto sia collocato presso la direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare, invece che presso l'ufficio legislativo. Il comma 2 aumenta da 19 a 21 il numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, in ragione dell'aumento dei componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate. Il comma in esame prevede inoltre che il legale rappresentante dell'impresa possa, in presenza di determinate condizioni, che sono state modificate durante l'esame in Commissione, assumere il ruolo di responsabile Infine esso inserisce le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato tra quelle che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che possono pertanto essere conferiti nei centri di raccolta urbani. La lettera *a-bis)*, introdotta durante l'esame in Commissione, disciplina, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio, un meccanismo di perequazione dei costi correlati agli obblighi di servizio

La Commissione ha introdotto il comma 3-*bis*, 60, cosiddetta legge Salva Mare, al fine di prevedere che i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti in plastica e in altri materiali accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, siano stabiliti ai sensi della disciplina generale contenuta nel codice dell'ambiente invece che da uno specifico decreto ministeriale. L'articolo 5 disciplina l'adozione del programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli incentivi degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova nonché, a seguito delle modifiche apportate in Commissione, dalle operazioni di drenaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara. L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, modifica la disciplina transitoria relativa ai valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica. proseguo nell'illustrazione del testo riprendendo dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di bonifiche finalizzate a consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di riqualificazione dei siti orfani. Il comma 1 reca disposizioni speciali per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, con particolare riferimento alla definizione del piano di caratterizzazione e all'approvazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica del progetto degli interventi. Il comma 2 dell'articolo 6 autorizza le Aziende regionali di protezione ambientale (ARPA) ad avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati, per lo svolgimento di una serie di analisi. Il comma 3 dell'articolo 6 apporta, infine, alcune modifiche al procedimento volto a determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni superino le soglie di contaminazione, nonché alla disciplina delle indagini svolte dalla Provincia per identificare il responsabile. L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale dovranno essere effettuati gli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara, istituisce la struttura di supporto del commissario straordinario e attribuisce a quest'ultimo un compenso aggiuntivo. L'articolo 8 reca disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo, in particolare sull'alimentazione del reparto nazionale degli interventi per la difesa del suolo, la piattaforma del e della banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso la Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico. Durante l'esame in Commissione è stato previsto che i piani speciali di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, in relazione alle aree colpite dagli interventi alluvionali del 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci che possono avere ad oggetto anche sole attività di progettazione. Si è poi previsto che le risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che siano state revocate perché non impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti e che siano state riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente siano impiegate dal segretario generale della stessa con i medesimi poteri e le medesime deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Sono stati infine stanziati 6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali. reca invece disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 prevede che, ai fini dello svolgimento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa adottare linee guida per settori specifici. I commi 2 e 3 dettano disposizioni in materia di determinazione del trattamento economico degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Il comma 4 autorizza il MASE a conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie ad assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR. Il comma 4-*bis,* introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che la maggiore impresa di trasporto del gas naturale partecipi, in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia, alla rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno, nelle more del recepimento della direttiva n. 1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno. Durante l'esame in Commissione è stato infine introdotto l'articolo 10-*bis,* recante modifiche alla disciplina dei finanziamenti che Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, tra l'altro, nel settore della tutela dell'ambiente e dell'approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche. Infine, l'articolo 11 prevede che dal decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 7 in materia di struttura di supporto e di trattamento economico del Commissario straordinario

molto problematici. Peraltro, lascio le considerazioni più generali alla senatrice Floridia Aurora, che parlerà più tardi o domani mattina (quando sarà) in dichiarazione di voto e potrà naturalmente fare un ragionamento più complessivo sulle ragioni per cui esprimeremo un dissenso nel merito molto forte e sulle ragioni per cui consideriamo questo decreto-legge molto poco a tutela dell'ambiente. Tuttavia, ho voluto anch'io intervenire in discussione generale per porre all'attenzione di quest'Assemblea qualcosa che è accaduto nel corso di questi giorni e di queste settimane e che, ahimè, potrebbe riaccadere nel corso dei prossimi giorni, essendo stata annunciata dal Governo,

della possibilità dell'ingresso di capitali privati nelle società che gestiscono l'acqua a livello comunale: le società *in house,* oggi a totale capitale pubblico. pubblico. Peraltro, ciò non è accaduto attraverso la presentazione di un disegno di legge organico, che perlomeno presenta un *iter* parlamentare, delle audizioni, una discussione, ma con un emendamento, che poi ieri è stato ritirato, probabilmente anche a seguito delle proteste inevitabili da parte delle opposizioni che ci sono state, per l'appunto in Commissione. Il Governo, però, ha già annunciato che lo ripresenterà, a quanto sembra, nella manovra finanziaria.

che queste destre, che si sono presentate in campagna elettorale due anni fa raccontando di se stesse come fossero una destra sociale,

è la più liberista delle scelte che si possano fare. *(Applausi)*. Peraltro, vorrei anche ricordare che questo emendamento 3.22, che per l'appunto apre la strada alla partecipazione dei soggetti privati nelle società a capitale pubblico, smentisce in maniera clamorosa il *referendum* che soltanto pochi anni fa aveva visto, in questo Paese, la stragrande maggioranza della popolazione italiana stabilire che l'acqua deve rimanere un bene comune, che l'acqua deve rimanere pubblica.

Divenne addirittura un momento di mobilitazione sociale e civile del Paese: il tema dell'acqua quale bene comune diventava davvero un valore attorno al quale costruire anche un momento di mobilitazione politica. Insomma, fu davvero un fatto straordinario, che accadde in Italia solo pochi anni fa. Ma davvero, dunque, si può pensare di stravolgere l'esito di quel *referendum* e immettere in un emendamento, ieri ritirato ma già annunciato per le settimane prossime, quello che rischia

dei servizi idrici nei Comuni? Io ritengo che ciò non si possa fare e quindi ho voluto e voglio così utilizzare questi minuti. Spero che lo facciano e sono certo che lo faranno anche le altre forze di opposizione,

vorrei dire anche con chiarezza di non cercare di sminuire la portata di questo emendamento, come pure è stato fatto in questi giorni. Gli elementi, che pure sono richiamati all'interno dell'emendamento e che le forze di maggioranza

invece non appaiono elementi sufficienti a giustificare la scelta che viene fatta dal Governo. È vero che si parla, testualmente: «della possibilità che il socio privato, direttamente o indirettamente, detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto», ma non può certo rassicurarci il fatto che soltanto il 20 per cento possa essere ceduto a un soggetto privato. Questo perché, evidentemente, anche una quota che non è maggioritaria può determinare un elemento assoluto di stravolgimento. Pensate anche alla storia degli anni passati. Il tema Il tema della privatizzazione non è qualcosa che si è inventata la destra italiana. Per questo io dico che questo è, per antonomasia, il più liberista dei temi possibili. La privatizzazione dell'acqua è stato il grande tema di battaglia politica che c'è che c'è stato, in particolare, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna una trentina d'anni fa, all'epoca dei Governi liberisti per eccellenza: quello inglese che faceva riferimento alla Thatcher e quello americano che faceva riferimento a Reagan. È lì che è nata la tesi secondo la quale bisognava andare a incidere sull'acqua e sulla gestione dell'acqua, ma sarebbe utile che andaste a vedere le conseguenze di quelle scelte. In quei Paesi, negli anni immediatamente successivi alla privatizzazione, aumentavano le tariffe e le bollette, ma peggioravano i servizi. Vogliamo allora davvero, anche in questo caso, fare finta di niente, smentire clamorosamente l'esito di un referendum e imitare i modelli che hanno funzionato di meno nel corso degli anni passati? Perché non provare invece a fare insieme quello che si sta facendo oggi in alcune grandi città europee, dov'è prevalente un modello radicalmente alternativo a questo, tutto centrato sul pubblico, come per esempio si fa a Barcellona o a Parigi, dove per l'appunto si cerca di mettere in campo un elemento d'innovazione, da una parte, che però salvaguarda il grande tema dell'acqua come bene comune,

quindi evidente e vero che esiste un grande tema che riguarda lo spreco dell'acqua, che non a caso, come tante altre cose in questo Paese, vede purtroppo un elemento particolarmente problematico al Sud. Davvero, però, qualcuno pensa che questa criticità si risolva con la privatizzazione, come se invece i modelli che sono stati inseguiti negli anni da altre parti non dimostrassero esattamente il contrario? Signor Presidente, lo dico ai relatori, al di là delle battute: questo intervento me lo sarei risparmiato, se nella giornata di ieri le forze di maggioranza avessero fatto la cosa giusta, cioè ritirare l'emendamento così com'era stato fatto; purtroppo però, nel momento esatto in cui lo ritiravano, comunicavano

spesso seguito dalla posizione della questione di fiducia, quindi il Parlamento è escluso dagli interventi emendativi in Aula. Ci resta quindi l'attività in Commissione, che - ora ve lo racconto - segue un *iter* alquanto peculiare, quantomeno nella mia esperienza diretta. Cosa accade? Quando ci troviamo di fronte a questa decretazione d'urgenza in seconda lettura al Senato, come abbiamo visto per il codice della strada, è stata introdotta a tutela della maggioranza, che vorrebbe intervenire su questi provvedimenti che evidentemente non reputa perfetti - la categoria degli ordini del giorno vincolanti, quindi un *escamotage* - il rito meloniano, direi - nella gestione di questi *iter*.

quella del sistema degli emendamenti accantonati. Si parte dal fascicolone degli emendamenti, il Governo dà i propri pareri (a parte le inammissibilità) e accantona

Si è arrivati così al ritiro da parte della maggioranza di un grande numero di emendamenti e chiaramente alla bocciatura di quelli dell'opposizione. Nonostante questo calvario e la fatica, l'opposizione non ha abbassato il livello dell'attenzione e nel fascicolo degli accantonati sopravvissuti anche all'ultimo setaccio abbiamo individuato un emendamento di Forza Italia che prevedeva - niente po' po' di meno - come già detto dal senatore che mi ha preceduto - la privatizzazione della gestione dell'acqua pubblica, con l'affidamento del servizio idrico ai privati. non era presente e, dopo qualche attimo di spaesamento tra le fila della maggioranza, un senatore coraggioso ha detto: lo faccio mio. A questo punto il Governo esprimeva parere favorevole. Chiaramente il MoVimento 5 Stelle, insieme a gran parte dell'opposizione, insorgeva con determinazione, richiamando gli esiti della consultazione referendaria che ha escluso che si possa fare profitto sull'acqua, che è un bene essenziale per la sopravvivenza e non può essere trattata e non può essere trattata alla stregua di una merce qualsiasi. Quindi, grazie ai nostri decisi interventi in Commissione, l'emendamento è stato prima nuovamente accantonato - e vabbè e poi ritirato dalla maggioranza, che è stata messa all'angolo da una contestazione sulla grande responsabilità di questa gestione. Per questa volta l'abbiamo scampata, ma non possiamo abbassare la guardia, perché questa insidia cova sotto la cenere. assistendo all'acutizzarsi dell'emergenza idrica, soprattutto nelle Regioni meridionali, dove ci sono milioni di italiani senza acqua.

La nostra risorsa idrica più preziosa è rappresentata dalle falde acquifere profonde, che purtroppo si stanno prosciugando. Queste sono le nostre riserve che ci possono garantire nel lungo periodo la disponibilità idrica. E perché mai si stanno prosciugando? Perché non percola nel terreno sufficiente acqua per ricaricarle a causa della gestione del territorio e della continua impermeabilizzazione del suolo. È proprio di ieri la presentazione del Rapporto annuale sul consumo di suolo che purtroppo ci dice che la tendenza non si sta invertendo. Paradossalmente, anche nelle aree dove ci sono problemi di dissesto idrogeologico (quindi nelle aree alluvionali) si continua a costruire, mettendo a rischio la sicurezza. Assistiamo quindi all'aumento delle impermeabilizzazioni e alla cementificazione e canalizzazione dei corsi d'acqua e, poi, il tutto viene condotto, con il cemento, a scaricare in mare. E come ricarichiamo di acqua dolce le nostre falde acquifere profonde se non lasciamo che l'acqua percoli attraverso il terreno? È chiaro che occorrono decenni perché le nostre casseforti d'acqua si ricarichino

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo provato a indirizzare l'azione governativa in questo senso. All'articolo 9 abbiamo chiesto interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, garantendo una quota del 20 per cento delle risorse per il recupero degli ecosistemi, anche nell'ottica dell'imminente attuazione della normativa *Nature restoration law*, che prevede, tra l'altro, il ripristino dei fiumi, delle acque e degli *habitat*. Sempre sull'articolo 9, siamo intervenuti sulle Grave di Ciano, dove si vogliono fare vasche di laminazione come opere di difesa idraulica del medio e basso corso del fiume Piave. Valutandone l'ambito territoriale, abbiamo chiesto l'alternativa ambientalmente meno impattante, perché le Grave di Ciano sono un sito protetto a livello europeo: Rete Natura 2000, Zona Speciale di Conservazione in relazione alla direttiva "Uccelli" e a tutto il Piano di gestione, Zona di Protezione Speciale. Quest'area non è a rischio idrogeologico, anzi prevede già naturalmente la possibilità di percolazione dell'acqua.

Abbiamo chiesto anche che venissero istituzionalizzati i cosiddetti contratti di fiume, che creano dei partenariati stabili, costituiti d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate. Abbiamo chiesto il finanziamento della Carta geologica d'Italia (Carg), perché, senza avere una previsione puntuale di come sta il nostro territorio, non riusciamo a programmare utilmente e a pianificare. Abbiamo chiesto che venisse riconosciuta l'impronta idrica, attraverso un'etichettatura ambientale, per identificare la *water footprint* nei prodotti commercializzati sul territorio nazionale, in modo che i consumatori possano avere contezza di quanta acqua viene consumata nel ciclo produttivo di quel prodotto. Abbiamo anche chiesto il riconoscimento dell'impronta del carbonio nell'ambito dei progetti di cui all'allegato 1-*bis* del codice ambientale, cioè i progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Quindi, proponiamo il criterio di selezione della *carbon footprint* del progetto tutto il suo ciclo di vita, garantendo un *fast-track* per i progetti più capaci di contribuire agli obiettivi energetici e climatici al 2030 e 2050, un criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi. Dopo tutto questo, ci è stato risposto

senza pensare alla salvaguardia degli ecosistemi, ammettendo nuove concessioni senza scadenza, perché è sino ad esaurimento dei giacimenti. Dovremmo arrivare a una decarbonizzazione con dei tempi fissati al 2030 e 2050, ma non si capisce bene come come si potrà raggiungere questo risultato. Dopo tutto questo balletto, tutte queste attese in Commissione, il Governo non ha avuto il tempo di approfondire, respinge tutti gli emendamenti e suggerisce: senatrice, presenti un ordine del giorno. Allora, per suo tramite Presidente, chiedo al senatore Rosso se questi ordini del giorno saranno considerati vincolanti come per il codice della strada.

oggi discutiamo di un provvedimento importantissimo che riguarda in maniera indiretta, attraverso la tutela dell'ambiente, anche la salute e la sicurezza della popolazione. È un tema fondamentale per qualunque territorio, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui più che mai l'ambiente è un'urgenza e una priorità, ma accanto ad esso si pongono anche diverse esigenze di sviluppo economico e di sicurezza energetica che vanno contemperate. Il decreto in discussione va a riformare per molti versi il testo unico ambientale del 2006, che ha rappresentato la prima riforma normativa organica in tema ambientale. Dal testo unico del 2006 sono tuttavia passati ormai quasi vent'anni ed è chiaro che da allora si sono poste, accanto all'esigenza della tutela ambientale, anche nuove esigenze parallele e oggi altrettanto pressanti, anche perché emerse abbastanza velocemente, soprattutto di recente con il precipitare di tutta una serie di eventi legati ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti geopolitici, alla sempre più agguerrita competitività internazionale sul piano della crescita economica, che si intersecano inevitabilmente anche con quella della tutela dell'ambiente. Esigenze nate cioè in un contesto economico in continua evoluzione che ha nella transizione energetica il suo punto cardine. cardine. Di fronte a queste nuove esigenze si è reso necessario intervenire sulla normativa. Ringrazio il Governo, in particolare il sottosegretario Gava soprattutto per il sostegno che ci ha sempre dato, per aver apportato con questo decreto una serie di modifiche sicuramente migliorative, in grado di dare

trova un fondamento unitario nella volontà di semplificare la normativa e velocizzare gli *iter* procedurali. Questo intento è perfettamente in linea con quella che è stata la politica della Lega da sempre e della maggioranza in generale, che ha sempre capito come una vera modernizzazione del Paese non possa che passare attraverso la sua sburocratizzazione. In questi mesi siamo stati chiamati ad affrontare sfide cruciali basate su impegni assunti dall'Italia a livello europeo e nazionale, in particolare attraverso il PNRR e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Per riuscire a vincere queste sfide e quindi a rispettare questi impegni indispensabile migliorare proprio l'efficienza e la velocità delle procedure amministrative che puntualmente rischiano di rallentare, se non bloccare, questi processi di sviluppo fondamentali. Questa velocizzazione, tuttavia, non deve travolgere e stravolgere altri valori, quali innanzitutto il rispetto dell'ambiente. Abbiamo quindi una serie di misure che si occupano di ambiente, ma contemporaneamente delle nuove emergenze connesse al cambiamento climatico, al dissesto idrogeologico, alla gestione delle risorse idriche e, non ultima, all'economia circolare. Difatti, il primo e fondamentale passo del decreto è un intervento sulle tematiche ambientali prioritarie, come le valutazioni ambientali, con previsioni che tentano di superare le criticità che hanno immobilizzato interi settori, come la coltivazione degli idrocarburi ma anche la messa in sicurezza dei territori e la bonifica dei siti contaminati,

l'economia circolare per limitare gli sprechi e promuovere la sostenibilità, miriamo a ridurre burocrazia e ritardi, che hanno finora ostacolato lo sviluppo dei progetti strategici, e offriamo importantissime opportunità di rilancio economico soprattutto alle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale In particolare, partendo dal primo articolo, acceleriamo le procedure di autorizzazione ambientale strategica attraverso modifiche sulle priorità dei progetti a cui le commissioni di valutazione ambientale devono dare precedenza per superare lo stallo in cui versano quelli che presentano maggiori complessità, e potenziamo le strutture delle Commissioni. Soprattutto, è importantissima l'introduzione del principio del silenzio-assenso, in mancanza di riscontro da parte delle Commissioni sulle richieste di sospensione del termine per presentare la documentazione integrativa da parte del Ministero della cultura sulla relazione paesaggistica presentata dal proponente. Sono tutte modifiche volte a garantire una maggiore rapidità nella realizzazione dei progetti ritenuti di rilevanza strategica. Ci occupiamo poi della sicurezza degli approvvigionamenti, con il divieto di rilasciare nuovi permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, però riducendo da dodici a nove dalla linea di costa e dalle aree protette il perimetro entro cui il divieto di svolgimento di queste attività. Anche qui viene contemperata l'esigenza di tutelare l'ambiente con quella dello sviluppo di un settore strategico per il Paese come quello energetico. Altre misure urgenti e necessarie di snellimento e razionalizzazione delle procedure sono poi introdotte in tema di siti contaminati, dissesto idrogeologico e crisi idrica. Partendo da quest'ultima, cito, tra le varie norme, quella che assegna nuovi compiti al commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, finalizzati al riutilizzo di quest'ultime. Riguardo alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, cito il potenziamento del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, con l'incremento del numero dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente interessate. l'intervento sugli scarti derivanti dalla cura e dalla manutenzione del verde pubblico e privato, la cui gestione viene oggi assimilata ai rifiuti domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di poterli conferire nei centri di raccolta urbani, facilitandone così l'operatività, oltre che la tutela ambientale. In tema di bonifica introduciamo, per esempio, misure speciali per consentire il raggiungimento entro le scadenze previste degli obiettivi del PNRR di riqualificazione dei cosiddetti siti orfani. Una norma, questa, a me particolarmente da senatrice del territorio calabrese. Fissiamo al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale dovranno essere effettuati

un ulteriore segno della sensibilità del Governo nei confronti delle popolazioni maggiormente colpite da scelte criminali in violazione dell'ambiente, ma anche della tutela della salute delle persone. Altro tema particolarmente grave e sentito è il dissesto idrogeologico. Anche di questo si occupa il decreto con una pluralità di norme profondamente innovatrici, che rispondono con estrema tempestività innanzitutto alle esigenze di chi è stato purtroppo pesantemente ferito dai danni dovuti al dissesto, ma anche di chi si trova in generale in aree a rischio. Vi è l'obbligo per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale di alimentare la piattaforma Rendis, a prescindere dalla fonte di finanziamento, per assicurare la completezza del quadro tecnico-conoscitivo, fondamentale per programmare e attuare interventi di prevenzione. Stabiliamo inoltre l'impignorabilità o il divieto di sequestro delle risorse finanziarie intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ai quali sono assegnate anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e che possono nominare appositi soggetti attuatori del Piano. Si tratta di un insieme di norme organiche e sfaccettate, che siamo certi potranno finalmente dare risposte serie ai territori. Torniamo ad occuparci dei disastri che hanno colpito Ischia, l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche, anche qui stanziando 10 milioni di euro per il 2024. Sono misure concrete che rinnovano l'impegno del Governo verso le popolazioni vessate da catastrofi climatiche e ambientali. Vorrei poi citare alcuni emendamenti che come Lega abbiamo portato avanti. Il primo è un emendamento che prevede uno stanziamento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2026 per reclutare e assumere personale presso le autorità di bacino distrettuali, superando una situazione di effettiva carenza di personale. Questo andrà a rafforzare la capacità operativa delle autorità di bacino. un altro emendamento che concede una proroga sui limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, consentendo alla filiera industriale, in modo particolare alle attività produttive che fino al giugno del 2022 avevano potuto usufruire della possibilità di conferire gli scarti non idonei al recupero presso siti di deposito definitivo, di poter continuare ad avvalersi dei limiti di accettabilità adeguati al volume dei rifiuti prodotti. Questa misura consente alle imprese di dare un sostegno anche dal punto di vista economico.

stabilendo i criteri e le modalità per la cessazione della loro qualifica di rifiuto. Tale misura dispone che i criteri saranno stabiliti con specifici decreti previsti a norma dell'articolo 184-*ter* del testo unico ambientale. Non siamo stati messi all'angolo come la senatrice prima sosteneva riguardo ad alcuni emendamenti che erano già stati accantonati dalla maggioranza e che poi sono stati ritirati perché necessitavano di ulteriori approfondimenti. La Commissione

la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico». Uno che legge questo titolo pensa che questo è un decreto-legge importantissimo e si darà un tempo sufficiente alle Camere per analizzarlo, trattandosi del bene ambientale che riguarda certamente le nostre generazioni, ma soprattutto le generazioni future,

Guardo con grande comprensione e solidarietà i tre moschettieri relatori che hanno difeso i loro emendamenti, devo dire senza successo, dalla bocciatura, il Presidente della Commissione e tutti i colleghi della maggioranza

che non si è trattato di un diniego motivato nel merito, perché c'è una politica diversa dal punto di vista ambientale, perché questo emendamento crea un problema con un'altra normativa o vogliamo fare un intervento successivo, successivo, ma perché in questo momento i decreti-legge servono per realizzare alcune questioni che dovrebbero essere urgenti al Ministro di turno e il passaggio parlamentare è un impiccio. Ci serve fare presto, andare veloci perché da questa parte del Parlamento, o da entrambe le parti del Parlamento, si perde soltanto tempo. Questo Governo

che vi chiede veramente e che purtroppo voi ancora esercitate: non la fiducia, ma la fedeltà, cioè l'adesione acritica ad una manifesta occupazione del potere, che non si capisce quale contenuto politico abbia. Non si tratta solo della frustrazione di membri del Parlamento dell'opposizione, ma anche della vostra frustrazione. Se voi non vi ribellate a questo meccanismo, a questo sistema, noi noi stiamo veramente facendo morire lentamente il Parlamento e, con il Parlamento, l'importanza del mandato che ci danno i cittadini. State facendo le prove generali di quell'idea di premierato che si basa su un'idea assoluta del potere di governo, che non è rispetto della libertà, ma esercizio di un arbitrio, cioè politiche economiche, regole e politiche ambientali senza un disegno complessivo. Noi avevamo presentato diversi emendamenti, per esempio su come potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico e alla siccità, soprattutto al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Guarda caso, ciò è avvenuto proprio nei giorni nei quali apprendiamo che il presidente della Regione Sicilia Schifani ha visto comunicare la cancellazione di 380 milioni di interventi per la Sicilia, perché evidentemente - sostengono - erano progetti

di questa istituzione, di cui è stato Presidente, ha capito che è di moda dire che è colpa dei Governi precedenti e quindi ci ha risposto così: la cancellazione di 380 milioni per la Sicilia è colpa dei Governi precedenti, solo che

di introdurre, all'interno del sistema di valutazione del cosiddetto ponte Salvini, la possibilità di un parere obbligatorio

ad un silenzio, cioè a quello che riguarda effettivamente i rischi ai quali vanno incontro i cittadini. Abbiamo inoltre proposto di risolvere una crisi industriale gravissima, che riguarda il polo industriale siciliano. In quel caso c'è una questione importante: il sequestro di un impianto di depurazione da parte della magistratura, a causa di DPCM sbagliati emanati da questo Governo, che hanno comportato la chiusura e il sequestro di un impianto di depurazione, che agisce e interferisce con un sito di interesse strategico per l'Italia, che porta il 32 per cento della raffinazione totale

che dell'ambiente, pare non se ne voglia occupare. Stiamo generando una crisi in Sicilia senza che questo Governo produca degli effetti, delle proposte, che risponda almeno alle nostre proposte, visto che noi continuiamo a farle, ma ci vengono bocciate. Nello stesso tempo abbiamo proposto di realizzare delle zone di interesse strategico nazionale, innovando sulla produzione produzione legislativa fatta in occasione del Governo Draghi dicendo qualcosa del tipo: visto che abbiamo dei siti di interesse strategico nazionale, proviamo a intervenire istituendo le zone di interesse strategico nazionale, che sono zone nelle quali esiste almeno un sito di interesse strategico nazionale, ma un ecosistema di imprese verso le quali possono essere attuate delle prescrizioni, se sono funzionali a mantenere vivo il sito nazionale di interesse strategico. In questo caso, ringrazio la Vice Ministra, perché l'emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno e su questo torneremo.

un soggetto privato che, anziché fare concorrenza nel mercato, avrebbe utilizzato la concorrenza per il controllo delle imprese, anche se, in questo caso, c'era un tetto alla partecipazione dei privati e di fatto avrebbe privilegiato discrezionalmente alcuni privati rispetto ad altri, al di là dell'evidenza pubblica della selezione, Questa è una cosa gravissima, perché di nuovo riguarda l'acqua, di nuovo riguarda un settore importantissimo che è in grande crisi in parti rilevanti del Paese. Ancora oggi, infatti, mentre io vi sto parlando, ci sono famiglie in Sicilia che non hanno l'acqua per uso civile e che devono pagare botti private per potersi rifornire. Abbiamo pezzi del PNRR che vedono cancellati questi investimenti in molte parti del Paese. Qui si è persa un'occasione importante, ma questo ormai lo ripetiamo da tempo. Ripetiamo da tempo che questo è un Governo che presenta, ogni volta, proposte di legge che rappresentano occasioni mancate. Siamo anche stanchi di ripetere che queste sono produzioni legislative di scarsa qualità. Sembra davvero un Governo a fine legislatura. Io non so se questo sia lo spirito con il quale pensavate di cambiare il Paese Sicuramente state offrendo uno spettacolo avvilente, non soltanto come Governo, ma a tutti noi. Noi chiediamo, a ciascun parlamentare della maggioranza, di avere un sussulto di orgoglio, di difendere voi stessi, di difendere noi stessi, di difendere la ragione per la quale siamo qui e per la quale siamo stati votati dai nostri cittadini. Siamo qui per cambiare le cose e non per dire semplicemente di sì, in silenzio, ad un esercizio di potere che è sempre più un arbitrio.

osservazione, una riflessione che mi è venuta ascoltando, in particolar modo, tutti gli interventi dell'opposizione e l'ultimo del collega Nicita. La maggior parte dei rilievi critici a questo provvedimento è stata fatta su una norma che non c'è, quella sulla presunta privatizzazione dell'acqua. Quindi, se le critiche a questo provvedimento sono su un emendamento che è stato ritirato e che non è presente nel provvedimento, vuol dire, evidentemente, o che i colleghi non avevano molti argomenti o che, come noi riteniamo, questo è un provvedimento positivo, utile, importante che, come già detto ampiamente dai relatori e dagli altri colleghi di maggioranza, va ad innovare, in modo anche sostanziale,

in questi due anni e poco più. Quindi è una tappa importante nel contesto di un lavoro su un tema che noi riteniamo assolutamente strategico e fondamentale. Vi sono norme, come è stato ricordato dai relatori, che hanno l'obiettivo di semplificare i procedimenti, in particolar modo sul tema dell'energia: semplificare, mettere chiarezza e fare ordine su una materia che è stata spesso oggetto, negli ultimi anni, di una grande confusione, anche normativa.

che hanno la possibilità di allacciarsi davvero a una rete di energia e che quindi sostanzialmente sono un contributo vero a una politica di energia basata anche sulle fonti rinnovabili, anche facendo cessare, come già abbiamo fatto con altri provvedimenti, un'azione meramente speculativa

Per affermare davvero - come noi pensiamo che sia possibile - una cultura dei rifiuti zero, che significa innanzitutto superare proprio il concetto di rifiuti, occorre lavorare a tutta la filiera, quindi sicuramente tramite la riduzione e il riuso, ma anche tramite l'attenzione alla realizzazione della filiera dell'impiantistica

vuole realizzare a Roma, perché in quel caso non si tratta di una chiusura del ciclo, ma di un ostacolo alla vera economia circolare. Occorrono quindi impianti con tecnologie moderne, che riducano le emissioni e siano finalizzati solo a tutto ciò che effettivamente non è possibile ridurre,

altrettanto importanti della messa in sicurezza del territorio e della cosiddetta questione climatica, anche qui, con concretezza e pragmatismo, nonché interventi effettivi che possano sostenere un territorio sicuramente fragile come il nostro, il nostro, al quale questo Governo sta dando molta attenzione, da questo punto di vista. È quindi necessario un rafforzamento delle autorità di bacino, anche con un intervento economico concreto di 6 milioni annui, per il potenziamento degli organici, al fine di dare la possibilità alle autorità stesse di fare interventi concreti sugli acquedotti e su tutto quello che può servire anche alla prevenzione rispetto al rischio idrogeologico. Vi è quindi, come dicevo, attenzione al territorio e alle comunità locali.

non significa però un'ecologia più blanda o una disattenzione al tema della tutela ambientale. Significa invece declinarla in un modo diverso, anche rispetto a quello che a livello nazionale ed europeo si è fatto prima dell'arrivo di questo Governo. Uomo e ambiente possono e devono coesistere, non secondo una visione di uomo separato, quasi dannoso e nemico dell'ambiente. Questo è stato

natura. In questo lavoro di custodia, allora, bisogna essere ovviamente proattivi, non osservatori come se si stesse in un museo ed è esattamente quello che noi stiamo cercando di fare. È quello che vogliamo fare, non solo ovviamente con questo provvedimento, ma con la nostra azione complessiva, diversamente da chi portava avanti una visione integralista, ma soprattutto dannosa per l'ambiente stesso. Ovviamente sto parlando della sinistra, soprattutto a livello europeo, ma anche nazionale. Quale beneficio c'è, c'è stato o ci sarebbe stato, ad esempio, a passare dalla dipendenza

(ricordiamolo sempre, casomai qualcuno se lo dimenticasse, visto che siamo nel tempio della democrazia) oltre a essere una dittatura, è soprattutto uno dei principali, se non il principale inquinatore del mondo. Quale convenienza ci sarebbe stata in una politica di questo tipo, che, tra le altre cose (lo stiamo vedendo in questi giorni), ha portato un contributo determinante nella crisi continentale e internazionale dell'*automotive*?

quello dei pannelli fotovoltaici. C'è chi voleva riempirne l'Italia, tra l'altro senza discernere, come invece noi abbiamo fatto con un altro atto normativo, le aree dove fosse opportuno realizzare

a come i pannelli, che ovviamente arriveranno presto a fine vita, dovessero essere smaltiti. Voglio ricordare che, grazie all'impegno di Fratelli d'Italia sia nella legge istitutiva della Commissione sul ciclo dei rifiuti, sia in un altro atto normativo che ha affidato al Gestore dei servizi energetici (GSE) alcuni compiti, risolveremo anche questo problema

Ci sentiamo assolutamente impegnati a portare avanti queste e tante altre politiche con un unico obiettivo, che è quello che ci ha lasciato in eredità un grande dell'ecologia, Paolo Colli,

Signora Presidente, dopo sette anni, che fanno 2.589 giorni di patibolo (non so come altro descrivere quell'agonia), le accuse pesanti rivolte a Stefano Esposito sono state finalmente archiviate. È demolito l'impianto accusatorio da un giudice non a Berlino, ma a Roma. Difficile dire che giustizia è stata fatta, perché dopo la sofferenza di questi anni, dopo il fango, il circo osceno delle polemiche, il lungo silenzio di chi "avrebbe dovuto esserci e invece", la battaglia che leva la pelle e l'anima per difendersi, è davvero impervio parlare di giustizia o di restituzione. In tutti questi anni, signora Presidente, Stefano Esposito non ha mai perso la sua dignità, certo non agli occhi della sua famiglia, al quale va il mio inutile e tardivo abbraccio, non agli occhi di chi si ostina a credere comunque nella giustizia, *contra spem*. Perché parlo di Stefano e della sua vicenda in quest'Aula? Per una impossibile abluzione autoassolutoria forse? Al contrario, se posso. Ne parlo innanzitutto perché Esposito è stato un senatore della Repubblica, due volte parlamentare, che ha servito con disciplina e onore il suo mandato e mi pare corretto che qui, proprio in quest'Aula che lo ha visto protagonista con la sua mercuriale generosità, con la sua ironia tagliente, con la sua passione civile, sia sottolineato questo giorno dopo tanta attesa, dopo troppo ingiusto tribolare. perché, Presidente, la sua assoluzione, alla fine della sua pena privata e pubblica (perché di pena si è trattato), è un atto di accusa. Parlo di noi qui, di un dibattito politico tra partiti che non possono tirarsi fuori e lo e lo vediamo in questi giorni di polemiche e scontri di nuovo attorno alla giustizia; nessuno è escluso da precise responsabilità sul fallimento di scelte e di riforme per evitare che questo succedesse - un innocente ingiustamente perseguitato - e che possa succedere ancora. un atto di accusa a comunità politiche, che spesso non sanno trovare, questa sì, la dignità del coraggio o il coraggio della dignità e farsi sentire presenti e non indifferenti, dalla parte delle garanzie che tutelano la vita di una Repubblica, dalla parte delle persone che finiscono schiacciate sotto una macchina implacabile che purtroppo conosciamo bene. E la nostra tepidezza e degnazione (parlo del Partito Democratico), l'onestà digrignata dei 5 Stelle, l'"in galera" della Lega e di Fratelli d'Italia, la cavillosità pelosa di Forza Italia, per fare nomi e cognomi - Presidente, me lo passi -, non è stata, non è temo e non sarà una risposta decente e utile alla domanda che ci pone questa storia, la sua storia, che è un po' anche una storia di questo Paese. Il senatore Stefano Esposito Il senatore Stefano Esposito - *semel abbas* - non è un caso. Il caso Esposito non è una grana, un incidente o una vittima designata. È un uomo che ha servito il suo Paese e questa Camera, non da, ma per il suo Paese, per questa Camera che lo ha accolto e aspetta ancora una giustizia che gli è stata ritardata

sul cibo ultra-processato, pubblicato in questi giorni da molte fonti di stampa. Per un totale di 19 milioni di decessi all'anno nel mondo sono 7.000 le morti al giorno causate dal consumo di alimenti trasformati, che portano problemi gastrointestinali, respiratori e cardiovascolari su tutto. Tale vera e propria carneficina conferma l'importanza delle nostre battaglie a tutela del *made in Italy* e del nostro sistema di eccellenza, con *standard* molto alti in tutte le fasi della produzione, come ci conferma il nostro modello alimentare fondato sulla dieta mediterranea, che ci permette, tra l'altro, di essere tra i Paesi più longevi al mondo. Il British Medical Journal evidenzia come gli alimenti trasformati creano una dipendenza più forte dell'alcol e del tabacco ed altre ricerche sottolineano anche come gli alimenti ultra-trasformati producano disturbi gravi alla salute. I cibi ultra-trasformati sono poi gli apripista per i cibi sintetici. Ricordo a quest'Aula che abbiamo approvato le norme che vietano la produzione e il commercio del cibo sintetico in Italia e le denominazioni ingannevoli attribuite ai prodotti trasformati. La Lega ha presentato anche un disegno di legge molto importante, a firma della collega Cantù, che riguarda il *rating* alimentare, che diventa fondamentale per stabilire la capacità di un prodotto di essere sano, genuino e capace di dare le giuste proteine alla persona. La Lega continuerà in ogni sede queste battaglie di buonsenso, soprattutto di trasparenza e di tutela di tutti i cittadini italiani. *(Applausi)*.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

la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"

Grazie